Onorevoli colleghi, come è a tutti noto, ieri sera la città di Strasburgo è divenuta il palcoscenico di un attacco omicida che, secondo un bilancio provvisorio, ha provocato la morte di almeno 3 persone e il ferimento di altre 13. Il nostro continente si ritrova a fronteggiare la volontà assassina di un terrorismo di difficile prevedibilità, in cui un singolo individuo può colpire persone innocenti in qualunque momento e in ogni luogo. Le istituzioni e le forze politiche devono individuare e attuare ogni strumento utile per contrastare la violenza prevaricatrice, al fine di difendere e preservare i valori di libertà e democrazia che costituiscono i fondamenti della convivenza europea. Proprio per questo è significativo come, pur nella drammaticità dei fatti di ieri, il Parlamento europeo abbia continuato la propria sessione dei lavori, dimostrando una fermezza che serve da esempio a tutti noi. Certa di interpretare il sentimento unanime della nostra Assemblea, rivolgo pertanto al presidente Antonio Tajani i sentimenti di profonda solidarietà. A nome mio personale e del Senato della Repubblica, esprimo la più stretta vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti e invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

degli articoli del disegno di legge «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».

In via preliminare si informa l'emiciclo che la Commissione giustizia, in sede referente, ha soppresso la lettera *r)* dell'articolo 1, comma 1, che era stata introdotta in Aula alla Camera mediante l'approvazione di un emendamento a scrutinio segreto, che derubricava alcune condotte relative al delitto di peculato inserendole nell'abuso d'ufficio. Passando in rassegna il provvedimento, esso si compone come segue. Il capo I interessa le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato, mentre il capo II è relativo alle misure in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Per quanto riguarda la relazione mi limiterò ad illustrare il contenuto delle disposizioni degli articoli da 1 a 8 del disegno di legge. in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, mirano in particolare a conformare l'ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di corruzione, a inasprire e ampliare l'ambito applicativo delle sanzioni accessorie, aumentare le pene e riformulare specifici reati, prevedere la collaborazione come speciale causa di non punibilità e introdurre nuove ipotesi di procedibilità d'ufficio, nonché ad apportare modifiche all'istituto della prescrizione. In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 aboliscono la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero da un cittadino italiano o straniero presente sul territorio nazionale, tramite l'introduzione di un nuovo comma agli articoli 9 e 10 del codice penale. La finalità di tali disposizioni è quella di adeguare il diritto interno agli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d'Europa. La lettera *c),* riformulando l'articolo 32-*quater* del codice penale, amplia il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (o comunque in relazione a essa), alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ai reati già previsti dall'articolo 32-*quater* sono aggiunti il peculato (escluso quello d'uso), la corruzione in atti giudiziari e il traffico di influenze illecite, come pure il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In conseguenza di ciò, la lettera *m)*, modificando l'articolo 317-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (perpetua o temporanea). La lettera *m)* integra il catalogo dei reati alla cui condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Infatti, agli attuali reati di peculato, concussione, corruzione propria e corruzione in atti giudiziari, la lettera *m)* aggiunge la corruzione impropria; la corruzione propria aggravata; l'induzione indebita a dare o promettere utilità; la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; la corruzione attiva; l'istigazione alla corruzione; i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri; il traffico di influenze illecite. Oltre all'indicato ampliamento del catalogo degli illeciti, è aumentata altresì la durata della misura accessoria temporanea, prevedendo un minimo di cinque e un massimo di sette anni in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a due anni, ove ricorra l'attenuante della particolare tenuità degli illeciti. Si prevede, invece, che l'interdizione temporanea sia compresa tra uno e cinque anni in caso di collaborazione, cioè quando il condannato si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. La lettera *d)* sostituisce il comma 1 dell'articolo 158, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato. La novità introdotta riguarda il termine di decorrenza per il reato continuato, fissato al giorno di cessazione della continuazione. Ulteriori rilevanti modifiche sono introdotte alla disciplina della sospensione della prescrizione. La lettera *e)* sostituisce infatti il comma 2 dell'articolo 159 del codice penale, stabilendo che, oltre alle ipotesi di cui al comma 1, il corso della prescrizione venga sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio, o alla data di irrevocabilità del citato decreto. Per finalità di coordinamento con le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione sono abrogati i commi 3 e 4 dello stesso articolo 159. Infine, la lettera *f)*, - anche in tal caso per esigenze di coordinamento con quanto previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo 159 abroga il comma 1 dell'articolo 160, che attualmente individua come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna. Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame individua nel 1° gennaio 2020 la data di entrata in vigore della disciplina della prescrizione, come introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale. Le lettere *g)* e *h)* - sempre nell'ottica di ampliamento e inasprimento delle sanzioni accessorie per reati contro la pubblica amministrazione introducono modifiche in materia di sospensione condizionale della pena. In particolare, la lettera *g)* modifica il comma 4 dell'articolo 165 del codice penale relativo agli obblighi del condannato per specifici reati contro la pubblica amministrazione che accede alla sospensione condizionale. Si tratta di disposizioni volte alla ripetizione del vantaggio indebitamente lucrato, che si collegano al contenuto dell'articolo 322-*quater*. La novella prevista

La lettera *h)* modifica invece l'articolo 166 del codice penale, relativo agli effetti della sospensione condizionale della pena, prevedendo che il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la pubblica amministrazione, possa disporre - in deroga alla regola generale - che la sospensione condizionale della pena non estenda gli effetti anche alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La lettera *i)* interviene sugli effetti della riabilitazione. A tal fine, si aggiunge un settimo comma all'articolo 179 del codice penale, che, derogando alla regola generale dell'articolo 178, stabilisce che la riabilitazione concessa sulla base della disciplina dello stesso articolo 179 non ha effetto sulle pene accessorie perpetue; prevede altresì la dichiarazione di estinzione della pena accessoria perpetua quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. La lettera *l)* integra il primo comma dell'articolo 316-*ter* del codice penale, aggiungendo un'aggravante del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, quando l'illecito è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri; in tali ipotesi, la pena è della reclusione da uno a Con la lettera *n)* sono inasprite le pene previste dall'articolo 318 del codice penale a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: è aumentata infatti la pena della reclusione sia nei limiti minimi (da uno a tre anni) che in quelli massimi (da sei a otto anni), con conseguente aumento anche dei termini di prescrizione del reato. La successiva lettera *o)* amplia l'ambito applicativo dell'articolo 322-*bis* del codice penale, che sanziona attualmente i reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Il disegno di legge, al primo comma, aggiunge due nuovi numeri che estendono la portata incriminatrice dell'articolo 322-*bis*: l'uno a carico di funzionari extra UE ovvero di chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale Una seconda modifica introdotta dalla lettera *o)* riguarda il secondo comma, n. 2), dello stesso articolo 322-*bis*. La novella amplia l'ambito applicativo della disposizione disposizione con riguardo ai funzionari esteri, eliminando l'elemento finalistico dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, di corruzione attiva e di istigazione alla corruzione. L'integrazione del contenuto della rubrica dell'articolo 322-*bis* del codice penale è infine dettata dalla necessità di coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera *l)* alla stessa disposizione. La lettera *p)* aggiunge al codice penale l'articolo 322-*ter*.1, con cui è stabilito che i beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contro la compresi tra gli articoli 314 e 320 del codice penale, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, nonché agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. La previsione è modellata sulla falsariga della custodia dei beni sequestrati nei procedimenti per reati tributari. Alcune modifiche sono state introdotte dalla lettera *q)* all'articolo 322-*quater* del codice penale, relativo alla riparazione pecuniaria conseguente a condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Anche in tale caso viene esteso l'obbligo del pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria anche al privato corruttore; viene soppresso il riferimento a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale; come anche viene stabilito che la somma da pagare da parte del condannato sia equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione lesa dalla condotta illecita.

una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria. In relazioni a questi fatti, caratterizzati da un accordo illecito, non è punibile colui che: li denuncia volontariamente; fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e gli altri responsabili. Per l'applicazione della causa di non punibilità occorre anche, però, che l'interessato sveli la commissione del fatto prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini in relazione a tali fatti

nonché disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. L'applicazione delle sanzioni previste, in base al nuovo assetto normativo, è posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, sia dei partiti sia dei movimenti politici. inoltre delegato alla definizione di un testo unico delle norme sulla materia. Nello specifico, l'articolo 9 reca norme in materia di trasparenza e controllo nei confronti dei partiti e movimenti politici. In particolare, al comma 1 si prevede un limite, fissato ad euro 500 annue per soggetto erogatore, sia che si tratti di somma di denaro o di prestazione o di altra forma di sostegno a carattere patrimoniale, quale contributo a movimenti politici

e per le liste e candidati alla carica di sindaco, che partecipino alle elezioni amministrative nei Comuni con più di 15.000 abitanti. Il primo consiste nella annotazione in un apposito registro, custodito presso la sede legale del partito o del movimento politico, di ogni forma di contribuzione ricevuta superiore, come valore, alla soglia dei 500 euro. L'annotazione deve essere realizzata entro un mese solare dal recepimento dell'apporto. Il secondo obbligo di pubblicità consiste nella pubblicazione, sul relativo sito Internet istituzionale del partito o del movimento politico ovvero della lista o candidato, del rendiconto contenente i dati sopra menzionati. È prevista un'esenzione dall'obbligo di pubblicità, ma permane l'obbligo del rilascio di ricevuta da parte del soggetto politico fruitore del servizio rispetto alle attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico. Al comma 2 viene espressamente fatto divieto, per i soggetti di cui sopra, di ricevere qualsiasi forma di sostegno proveniente da soggetti giuridici esteri, qualunque essi siano. È inoltre introdotto il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto, di elargire contributi a partiti o movimenti politici, ovvero alle liste e ai candidati che partecipino alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti. Il comma 3 prevede che i contributi ricevuti in violazione degli obblighi di pubblicità o dei divieti previsti non siano ripetibili e debbano essere versati alla cassa delle ammende. Il comma 4 dispone che entro il quattordicesimo giorno antecedente lo svolgimento di qualsiasi competizione elettorale, ad eccezione dei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste che si presentano alle amministrative dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet il *curriculum* e il certificato penale dei candidati. In questo modo viene consentito all'elettore un facile accesso alle informazioni. Il comma 5 specifica che la pubblicazione dei predetti documenti debba avvenire presso il sito Internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno nel caso di elezione politiche o europee, presso apposita sezione denominata: "Elezioni trasparenti". Il comma 6 istituisce un obbligo di trasmissione relativo ai rendiconti e i relativi allegati alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei partiti e movimenti politici. L'articolo 10 interviene, a integrazione e completamento rispetto a quanto già disposto dall'articolo precedente, con diverse modifiche alla normativa vigente in materia di pubblicità e tracciabilità dei contributi erogati verso partiti politici e soggetti titolari di cariche elettive e di Governo. Più nello specifico, il comma 1 modifica in più parti il vigente articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013 (abolizione del finanziamento pubblico ai partiti). La modifica introdotta dalla lettera *a)* riduce da 5.000 a 500 euro il limite dell'importo annuo ricevuto a titolo di liberalità da parte dei soggetti titolari di cariche elettive e di Governo, ivi inclusi i tesorieri dei partiti, sopra i quali vi è l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto direttamente o attraverso i comitati di sostegno. La lettera *b)* del comma 1 sopprime il comma 3 del vigente articolo 5 del citato decreto-legge n. 149 del 2013. Gli articoli 11 e 14 recano disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti fra partiti, movimenti e fondazioni politiche. In particolare, l'articolo 11 prevede che gli obblighi di trasparenza e rendicontazione in capo a partiti e movimenti politici siano applicati ad associazioni, fondazioni e comitati, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazione di partiti o movimenti politici, ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero da persone che siano o siano state nei dieci anni precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che ricoprano, o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, ovvero incarichi istituzionali per essere stati eletti o nominati

recante un testo unico a scopo di coordinamento normativo fra le varie disposizioni. L'articolo 12 reca le sanzioni amministrative pecuniarie susseguenti alle violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo. L'applicazione della sanzione compete alla Commissione per la trasparenza. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni saranno versate alla cassa delle ammende.

spazza corruzione, ma che oggettivamente spazza ben altro, ovvero i principi elementari del nostro sistema giudiziario. Preliminarmente, occorre sottolineare la disponibilità che il Partito Democratico ha manifestato nell'affrontare il percorso di questo disegno di legge, con spirito aperto, costruttivo, partecipando all'*iter* del provvedimento sia alla Camera che al Senato. Ebbene, tutto questo è avvenuto in maniera del tutto inutile. Una volta giunto presso questo ramo del Parlamento, la situazione è anche peggiorata - se possibile - in quanto il testo ha subìto una sola modifica per porre rimedio a quella trappola che era stata fatta evidentemente da qualcuno della stessa maggioranza, considerati i numeri,

La discussione presso la Commissione giustizia - è triste doverlo dire - è stata del tutto irrispettosa di qualunque prerogativa dell'opposizione, con una maggioranza sorda a qualunque richiesta e a qualsivoglia confronto nel merito del testo e delle disposizioni più critiche che presenta. Eppure il Partito Democratico, come già è stato evidenziato anche in Commissione e in precedenza, ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo e responsabile perché è consapevole che la lotta alla corruzione e all'illegalità che si annida nella pubblica amministrazione costituisce una necessità, un obiettivo inesausto della politica in un Paese come il nostro nel quale il fenomeno è ancora tristemente endemico e diffuso. Lo abbiamo fatto perché nel corso della XVII legislatura la lotta alla corruzione è stata la priorità di tutti i Governi a guida del Partito Democratico. Si pensi alla legge n. 69 del 27 maggio 2015 - l'anticorruzione del 2015 - che ha inasprito le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, ha reintrodotto il falso in bilancio che era stato cancellato, ha subordinato la concessione della sospensione condizionale alla restituzione del maltolto. pensiamo all'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio, all'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione che benissimo funziona e che è dotata del personale e delle risorse per operare, al reato di scambio politico-mafioso e, non da ultimo, all'introduzione di quella che era sostanzialmente la denuncia delle violazioni da parte di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione stessa con la previsione della tutela dagli atti ritorsivi nei confronti delle persone che segnalavano questi questi fatti. Devo dire che questa era stata un'iniziativa dell'opposizione che aveva trovato, però, ampia collaborazione da parte dell'allora maggioranza, il che aveva consentito di approvare un testo che è estremamente importante nel nostro sistema. Il testo che quest'Aula si trova oggi ad esaminare suscita rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Anzitutto non si può tacere la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che modifica diversi articoli del codice penale. Entrando nel merito, all'articolo 166 del codice penale è aggiunta la previsione in base alla quale per alcuni reati, diversi tra di loro, il giudice possa disporre che la sospensione non estende i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. A tale riguardo, si rileva che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die* in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese l'articolo 3 della Costituzione, ma questo, ovviamente, sarà oggetto della discussione che avverrà nel corso dell'esame degli emendamenti e quindi non intendo dilungarmi perché di altre cose ben più importanti bisogna parlare. Venendo al merito della riforma introdotta si rileva anche l'introduzione del tema della prescrizione. Ora, si rileva come la prescrizione sia un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune nonché soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale in quanto si lega alla sentenza n. 393 del 23 novembre 2006. La natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, prima fra tutti la collocazione dell'istituto, non a caso, nel codice penale. Pertanto la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione e dunque le scelte del termine prescrizionale sulla sua disciplina sono da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali, prime fra tutte, com'è noto, il rispetto dell'articolo 111 della Costituzione che prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi, per l'appunto, ragionevoli. Oggi, sostanzialmente, in questa maniera si violano i diritti di tutte le parti del processo. L'imputato, con l'introduzione di questo nuovo sistema della prescrizione, corre il rischio di vedere un processo che si allunga a dismisura. La parte civile, la parte offesa, non potrà vedere riconosciuti i suoi diritti perché sicuramente i processi si allungheranno notevolmente nel tempo perché conosciamo lo stato degli uffici giudiziari. Si ricorre ad un sistema che non è sicuramente utile se si considera che, per i dati che ci sono stati forniti dallo stesso Ministero,

una piccolissima osservazione, visto che viene introdotto in questo provvedimento che si occupa di anticorruzione: i reati che si prescrivono relativi ai ai delitti contro la pubblica amministrazione sono una parte minimale, equivalente a circa il 3-4 per cento del totale, una parte bassissima. Conseguentemente non si avrà alcun risultato effettivo. Ma ancora una volta questa maggioranza vuole semplicemente fare provvedimenti *spot* che di fatto non portano Altra cosa sarebbe stata se si fosse introdotto un nuovo sistema, se si fossero previsti metodi per evitare le prescrizioni, rafforzando il sistema giudiziario con la previsione di un numero sufficiente di giudici che consenta finalmente di avere un organico pieno, una magistratura togata anziché affidarsi come sempre alla magistratura onoraria (come sta accadendo ormai da troppo tempo),

modo, ci si dica perché non si rafforza il personale amministrativo, che consentirebbe immediatamente di dare una risposta seria ed evitare che molti processi vadano prescritti. prescritti. È anche necessario ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 31 maggio 2018: «La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno…». È evidente che il problema della prescrizione esiste, ma i sistemi per combatterla solo quelli di cui ho parlato in precedenza. Ancora, di analoga gravità appare anche la novella dell'articolo 179 del codice penale, che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione. Anche questi sono provvedimenti palesemente incostituzionali.

Qui si è detto che non si tratta di agente provocatore, ma di infiltrato. Leggete il testo - ne parleremo quando arriveremo all'esame degli articoli - e vi renderete conto che non di infiltrato si tratta, ma di agente provocatore vero e proprio. Ripeto, basta leggere il testo: è evidente che si tratta di agente provocatore. A questo riguardo, voglio ricordare anche che le direttive europee vietano in maniera nettissima e ferma che si possa far ricorso all'agente provocatore nei reati contro la pubblica amministrazione. Non di meno, anche questo viene previsto, insensibili a qualsiasi indicazione che ci viene dall'Europa e dalla nostra Costituzione. In conclusione, signor Presidente, noi consapevolmente affermiamo che si tratta ancora una volta di un provvedimento *spot*, un provvedimento *spot*, privo di vero contenuto riformatore. Noi avevamo già dato una riposta seria, che sta funzionando nella lotta alla corruzione con i provvedimenti di cui ho parlato e che - lo ribadisco - erano stati approvati nella scorsa legislatura con la massima collaborazione tra le forze di maggioranza e di opposizione. esame - lo ribadisco - è infarcito di norme di dubbia costituzionalità e sarà verosimilmente approvato, ancora una volta, senza alcun confronto serio e costruttivo, senza alcun dialogo tra le forze presenti in quest'Aula e sarà approvato esclusivamente, per l'ennesima volta, con la sola logica dei numeri, e questo ovviamente non è un metodo che può andar bene in un sistema democratico come il nostro.

una relazione di minoranza e la risposta è stata positiva, perché l'*iter* legislativo di questo disegno di legge pone una serie di problemi sulla tenuta del nostro sistema democratico. Mi riferisco al fatto che, mentre alla Camera dei deputati abbiamo avuto un ampio ricorso alle audizioni di esperti e tempi di discussione accettabili sia in Commissione che in Aula, il disegno di legge perviene al Senato per la semplice abrogazione di un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, con una singolare interpretazione del bicameralismo e della possibilità di approfondimenti che la Costituzione assegna a ciascuna delle Camere. È stata negata la possibilità di effettuare audizioni in questo ramo del Parlamento e la discussione ha registrato solo interventi e emendamenti dell'opposizione, fatta eccezione per l'emendamento abrogativo preteso da una parte della maggioranza, perché il testo approvato non era stato concordato dalle due componenti del Governo. Tale situazione pone non pochi interrogativi, primo tra tutti la conclusione che si può trarre da tale comportamento: il Parlamento, per l'attuale maggioranza, è inteso come mero esecutore del volere del Governo, per cui un emendamento approvato con libera determinazione della Camera dei deputati deve essere eliminato e al più presto, senza alcuna possibilità di discutere ed esaminare le altre norme del disegno di legge. È questo il bicameralismo per il quale ci siamo battuti insieme durante il *referendum* costituzionale? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. E voi, partiti della maggioranza, allora avevate bene inteso qual era il ruolo che spetta a ciascuna delle Camere e qual era il ruolo dei partiti politici. È forse utile che in quest'Assemblea, signor Presidente, si organizzi un dibattito sui princìpi della nostra Costituzione e sulla democrazia parlamentare che è un effetto della democrazia rappresentativa. Certamente invece una riflessione va fatta - ed è necessaria - sul nostro Regolamento, che nel prevedere il tempo di dieci minuti, non tiene conto dell'importanza di alcuni articoli, come l'articolo 1 del disegno di legge in discussione

a una conseguenza necessaria: i cittadini non hanno la possibilità (perché non viene loro consentito) di comprendere a fondo non solo le ragioni delle tesi della minoranza, minoranza, ma nemmeno le motivazioni che sorreggono la norma proposta dalla maggioranza, specie se - come è avvenuto - a fronte di dati statistici che avrebbero giustificato quantomeno una riflessione, il silenzio della maggioranza e l'assenza di qualsiasi confronto generano la sensazione dell'inutilità dell'attività parlamentare. La sfiducia dei cittadini nella politica - e a tratti nelle istituzioni - non può essere alimentata da norme e comportamenti relativi all'attività parlamentare. il disegno di legge introduce molteplici modifiche di diritto sostanziale e processuale, che in gran parte si pongono in contrasto con la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale.

in contrasto con il sistema giudiziario del nostro Paese. Ciò ha determinato la critica - come avete visto - non solo degli avvocati, ma anche dei magistrati e di tutti i giuristi; nessuno di quelli che avete audito alla Camera vi ha dato un minimo di spazio di ragione. Può dirsi infatti accettata nel nostro Paese la teoria del doppio binario e cioè un trattamento eccezionale riservato ai reati di particolare gravità, come mafia e terrorismo, e che si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e di interdizione, nonché a sanzioni particolarmente elevate, e uno, invece, per così dire ordinario, per il quale sono irrinunciabili le garanzie che nel primo binario sono compresse per esigenze di difesa sociale. Che i reati contro la pubblica amministrazione, pur destando un elevato allarme sociale, possano essere considerati sullo stesso piano dei reati di stampo mafioso o camorristico è fuori da qualsiasi logica. Non vi è alcun dubbio che non c'è paragone possibile tra mafia e terrorismo e questi reati, in particolare perché non sono comparabili con fattispecie così gravi perché le statistiche confermano che l'accertamento giudiziario dei reati contro la pubblica amministrazione è più che soddisfacente, con tassi di prescrizione del tutto irrilevanti. Se volete discutere - ma non siete abituati a farlo - sulla base dei dati, dovete riconoscere che nel nostro Paese non esiste attività delittuosa contro la pubblica amministrazione che non venga perseguita. È ridicolo, infatti, pensare che i fenomeni corruttivi siano di gran lunga superiori a quelli accertati: non ha alcun fondamento,

degli indizi rilevanti di fattispecie penali rivelatisi insufficienti o non idonei a contrastare un fenomeno, oppure interviene con nuove norme e nuove fattispecie di reati, quando i nuovi comportamenti antigiuridici non risultano avere una rilevanza penale. Questo non è avvenuto. Non abbiamo alcun elemento per dire che i reati contro la pubblica amministrazione non siano perseguiti nel nostro Paese con tutta le garanzie, ma, nello stesso tempo, con tutta la durezza che quei reati necessitano sia applicata da parte dello Stato. I dati statistici, non inventati dalla minoranza, ma forniti dal Ministero della giustizia, se letti correttamente, evidenziano non solo che l'indice di prescrizione di questi reati

Ma vi rendete conto di quanto sia ridicola questa affermazione? La corruzione viene scoperta tardi, però la prescrizione è bassa. Se fosse così, la prescrizione per reati contro la pubblica amministrazione perché, scoprendosi tardi, non ci sarebbe il tempo per la celebrazione del processo. Si deve, ancora, tener conto che per tali reati il tempo necessario a prescrivere è già estremamente lungo.

i dati forniti dal Ministero dimostrano che la prescrizione è diminuita ogni anno. Addirittura in alcuni tribunali e in alcuni uffici la prescrizione è quasi pari a zero. Se allora il Ministro della giustizia, anziché presentare una norma che non aveva nulla a che fare con questo disegno di legge, avesse dato un minimo di attenzione ai suoi dati, avrebbe capito che in alcuni uffici giudiziari la mancanza di strutture e di organici ha determinato quelle prescrizioni che negli altri uffici non si verificano. per cento dei tribunali italiani non ha prescrizioni. Questa riforma porterà all'allungamento dei tempi di tutti i processi,

Vi rendete conto che questa non è un affermazione, ma è una rilevazione basata sui dati forniti dal Ministero?

diminuzione di 57,2 miliardi alla giustizia e indovinate per che cosa? Per la riforma del processo penale

C'è poi una situazione di contrasto con i princìpi costituzionali per quanto riguarda tutto ciò che inerisce alle pene accessorie. vi rendete conto che significa non capire nulla di diritto penale generale pensare che una pena accessoria possa durare in eterno rispetto alla pena principale.

nei princìpi della nostra Costituzione, in base ai quali ciascun cittadino, responsabile e colpevole di qualsiasi reato, ha la necessità di essere rispettato e di avere la possibilità di redimersi. Se non ci fosse questa *chance*, se non ci fosse questa possibilità per l'imputato di redimersi, non avrei fatto il magistrato.

non so se mi basteranno cinque minuti, perché ieri sera mi sono messa a fare l'elenco degli articoli della Costituzione che questa normativa che andiamo ad approvare viola

quello relativo al principio di uguaglianza, quello relativo al principio di colpevolezza, quello relativo alla libertà economica

Non mi rivolgo al Governo, perché ritengo che il Governo non meriti neanche un'interlocuzione da questo punto di vista. Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega, che hanno mandato avanti questo provvedimento in Commissione in una sorta di marcia a tappe forzate: lo abbiamo approvato all'una di notte, in una nottata. nottata. Se oggi andrete ad approvare questo provvedimento e non lo bloccate con la questione pregiudiziale, approverete una normativa per cui sulle vostre personali coscienze ci saranno famiglie distrutte, eterni eterni innocenti che aspettano un giudizio, gente che va in carcere perché diventano tutti reati ostativi, e ci saranno persone, magari vittime di errori giudiziari, che non vedranno mai la luce.

ha la cattiveria sociale che si esprime con il provvedimento al nostro esame e non è tutelato dai provvedimenti, come ricordava il senatore Caliendo, relativi al bilancio. Ci troviamo semplicemente di fronte a un un provvedimento che dice «sei incappato per caso nella giustizia dei reati contro la pubblica amministrazione, va bene, rimani dentro, chiudo con la chiave e di te non ne voglio sapere più niente».

Se infatti le persone sono in condizioni di cattiveria, lo sono perché non hanno i soldi per arrivare a fine mese e non perché vogliono vedere

ha proposto una serie di emendamenti migliorativi, perché ha sempre mantenuto la linea dettata ed esplicata dal Presidente del Gruppo, ribadendo che noi siamo un'opposizione comunque costruttiva. Si trattava di emendamenti

non solo il fantomatico colletto bianco che vogliamo vedere in galera perché così diamo sfogo alla cattiveria sociale: è di questo Abbiamo ancora il caso di un cancelliere che è stato condannato in terzo grado per peculato perché si era appropriato di un contributo unificato di 35 euro.

affossa il mondo produttivo, perché colpisce non solo il soggetto colpevole, da un punto di vista personale, ma mette una croce sopra all'attività d'impresa. Ci sono imprese imprese che sono saltate nel nostro Paese proprio perché i pm hanno disposto sequestri di quote e voi così date loro la mano libera di affossarle: ve l'hanno detto gli industriali alla Camera a chiare note. L'associazione che fa l'indicizzazione della corruzione vi ha anche detto - per i partiti politici, perché anche lì si va a ledere la base dell'articolo la base dell'articolo 49 della Costituzione - che questa roba così strutturata non è applicabile, perché non abbiamo una normativa sulle *lobby*. Questo l'ha detto

dettata dalla cattiveria sociale e alla quale tutto il mondo del diritto vi ha avvertito di prestare attenzione. Ma tanto voi non ascoltate: fate i tavoli quando siete con l'acqua alla gola, con un Ministro che convoca qualcuno di qua e

forte. Avrete sulla coscienza le persone che finiranno sotto questa normativa, fatta solo per dimostrare che due *leader* hanno i numeri in Parlamento: li avrete sulla coscienza per tutta la vita.

la prima osservazione che sorge è che a nessuno di questa maggioranza di Governo viene negata la sua norma manifesto. A ciascuno la sua ed eccoci di nuovo alle norme manifesto. È particolarmente importante sottolinearlo quando valutiamo la compatibilità con i princìpi costituzionali

Questo è grave, soprattutto da parte di chi in altre occasioni ha imbracciato la Costituzione, ma probabilmente l'ha rimessa nel cassetto, chiudendola a doppia mandata.

sarà l'ultima) ha in comune il fatto di rappresentarsi una diversa idea o forse un capovolgimento dello Stato di diritto,

provvedimento in titolo, del quale non vi era bisogno se non per affermare il principio del superamento dello Stato di diritto e della democrazia liberale, perché le norme sulla corruzione sono state approvate recentemente e perché, come è stato detto, per

e l'efficacia del processo, perché quando si prevede una durata *sine die* del processo, sostanzialmente si sta celebrando la sua irrilevanza. Non c'è alcun intervento per rendere efficace il processo.

violazione del principio di uguaglianza, perché vengono disciplinate in modo uguale situazioni diverse, irragionevolezza in una pena accessoria *sine die* che addirittura addirittura non viene recuperata con la riabilitazione e non è coperta dalla sospensione condizionale della pena. Quando parliamo di riabilitazione intendiamo reinserimento, recupero della persona condannata, condannata, restituzione alla collettività di persone migliori, attività di restituzione senza le quali la riabilitazione non viene concessa.

che consistono in assegnazione al lavoro esterno, permessi premio, misure alternative; stiamo discutendo del fatto che una persona condannata per questi reati non possa e non debba

fronte all'idea che punire impedendo di lavorare possa evitare la corruzione e possa mettere sulla pubblica piazza qualcuno da indicare. Qui non siamo al processo: qui siamo al pollice verso dei riti che si celebravano al Colosseo. E che dire dell'agente provocatore (perché di questo si tratta)? È una questione

Quando parliamo di condotte nei reati di corruzione, ci riferiamo a un reato a concorso necessario. Stiamo parlando di un reato che si basa sull'allettamento, sull'invito a, su una serie di condotte, zone grigie e inviti a infrangere la legge. Dove è il principio di legalità?

quando si invocano pene più severe - e l'abbiamo fatto - quando si invoca l'efficacia delle decisioni - e l'abbiamo fatto - quando si invoca il fatto che i reati di corruzione, certo, destano scandalo e vanno puniti,

la legalità nell'allettare e invitare a infrangere la legge (perché questo è l'agente provocatore). Per saggiare cosa? Un livello etico di cui si smarriscono i confini, perché chi rappresenta la legge invita a infrangerla. Mi avvio

quando si pronuncia una sentenza in nome del popolo italiano è un momento di controllo pubblico e democratico del rispetto della legalità. Un processo senza fine, che danneggia non solo chi è accusato, ma - soprattutto - le vittime dei

creiamo, modifichiamo e interveniamo sui reati, al fine di ottenere giustizia, per fare in modo che i reati vengano perseguiti e possano esserci pene efficaci, perché applicate in tempi rapidi e visibili a tutti.

delle gravi criticità: non lo nascondiamo e, anzi, lo affermiamo con decisione. Condividiamo molte delle perplessità e delle critiche contenute nelle questioni

rendiamo il servizio che siamo chiamati a svolgere in quest'Aula per migliorare i provvedimenti che vengono presentati e per dare alla società civile e all'Italia la giusta risposta contro la corruzione, che è un veleno che distrugge i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, è un veleno che distrugge la libera concorrenza, è un male che noi vogliamo contribuire a combattere.

Non siamo pertanto d'accordo con la riforma della prescrizione; entreremo nel merito quando sarà il momento, ma già ora diciamo che riteniamo questa riforma della prescrizione palesemente incostituzionale. Essa viola il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione, viola l'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, viola gli stessi diritti delle persone offese, parte civile, che vedono procrastinato all'infinito il loro giusto diritto a una pronuncia, viola il il diritto dell'imputato, che, fino a prova contraria, deve essere considerato non colpevole e che invece si vede condannato a un processo senza fine, che diventa la vera pena. Ci sono poi molte altre ragioni, che illustreremo in sede di discussione generale. Così come siamo molto preoccupati per la previsione di cui all'articolo 6 di questo disegno di legge che, pur chiamandolo agente sotto copertura, in realtà introduce un vero e proprio agente provocatore, dichiarando non punibili persino le attività prodromiche prodromiche e preparatorie e persino la promessa della dazione di danaro, da parte di colui che non è più quindi un agente infiltrato, ma è un vero e proprio agente provocatore. Per queste ragioni, cari colleghi, noi ci asterremo nel voto sulle pregiudiziali, non perché non condividiamo molte delle perplessità manifestate nelle pregiudiziali stesse, ma perché abbiamo fiducia, nonostante tutto, che il Senato, entrando nel merito delle questioni, saprà dare la giusta risposta.

vi spiegherò per quale motivo il mio Gruppo e in particolare i senatori del Partito Democratico chiederanno a tutti gli altri colleghi di votare a favore di questa pregiudiziale di costituzionalità. La Costituzione è continuamente evocata in tutti i vostri ragionamenti propagandistici. Nella scorsa legislatura, la XVII, con infinito impegno e dedizione avevamo provato a portare avanti un lavoro di modifica ma nel pieno rispetto della Costituzione, mentre voi, che tanto sbandierate il fatto di aver resistito, nella scorsa legislatura, a questo lavoro di modifica, adesso fate stralcio continuo, come un fazzoletto con cui vi soffiate il naso, di tutto ciò che la Costituzione prevede. pregiudiziale cerchiamo di spiegare, come ha fatto prima di me la collega Rossomando (ma mi richiamo anche all'intervento svolto in Commissione giustizia dalla senatrice Modena), che in questo testo voi affermate solo ed esclusivamente la logica della vendetta, la logica della vendetta che si ispira all'odio sociale, la logica della vendetta del fine pena mai, perché introducete il fine pena mai nelle pene accessorie anche davanti a casi di assoluzione. Voi avete abituato l'Italia, avete abituato gli italiani, una parte degli italiani, parlando alla loro pancia, a una gogna mediatica infinita. E, guardate, fate male a parlare di giornali, giornalini e giornaloni, perché la gogna mediatica l'avete inventata voi, in quello schifo di sacro *blog* nel quale additate le persone, le mettete alla berlina, chiedete che ci siano continui richiami («condividete!», «condividiamo!»), esportate E adesso lo volete fare all'interno del processo penale. Cercheremo di non consentirvelo, perché non è questo il modo di trattare né la Costituzione, né il luogo più alto delle garanzie costituzionali, che è proprio il processo penale.

l'articolo 111 della Costituzione, che richiama il giusto processo. L'ha detto bene un attimo fa, prima di me, il collega Balboni, con il quale non condivido proprio nulla, ma in realtà anche lui, nella sua attività

sono tutte quelle persone che sicuramente attendono la condanna, ma attendono, per esempio, anche un risarcimento. Non è un caso che la maggioranza dei processi in questo Paese si prescriva ancora nella fase dell'indagine preliminare, dove molto spesso ancora non c'è la costituzione di parte civile, perché, come sanno anche i nostri allievi del primo anno di giurisprudenza alla Sapienza, ci si può costituire entro la prima seduta seduta di udienza dibattimentale o nell'udienza davanti al gup. Quindi date anche uno schiaffo alle vittime.

proprio per la dubbia legittimità costituzionale del primo articolo di questo scellerato disegno di legge, che, andando a modificare l'articolo 166 del codice penale prevede che, per alcuni reati, anche diversi tra di loro, anche con condotte diverse e con diverse fattispecie, quindi con comportamenti di gravità diversa, il giudice possa disporre che «la sospensione

il principio più sacro, quello dell'uguaglianza tra tutti i cittadini, e che a me personalmente sta più a cuore quando si parla di diritti delle persone. Voteremo a favore della questione pregiudiziale che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die* in maniera fissa, senza gradualità e ben oltre la durata della pena principale, viola tale articolo in modo aperto. Voteremo sì alla questione pregiudiziale, perché l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costituzionale di uguaglianza, finendo per trattare in modo uguale situazioni molto diverse tra di loro. Quindi, questa disposizione, a nostro parere, appare difficilmente conciliabile

quest'anno, non datata, ma fresca, nuova. La Corte ribadisce che il legislatore è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata; resta una facoltà del legislatore, in particolare, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati. Tuttavia - sottolinea il giudice delle leggi nella medesima sentenza - la discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza. Il principio di ragionevolezza, colleghi, è presente nell'articolo 111 della Costituzione e prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi ragionevoli,

perdere le tracce di quello che è accaduto, non avere neanche la citazione per una minima raccolta di prova o di incidente probatorio del proprio avvocato, e magari leggere dopo sei mesi, dopo uno o due anni che quell'indagine è ancora in corso perché magari una velina è arrivata a un giornale, guarda caso, nemico forse di quel parlamentare o di quel sindaco. Voglio aprire una riflessione su questo: attenzione, perché proprio voi, nel vostro sacro *blog*, additate spesso i nostri sindaci, i nostri consiglieri regionali, i consiglieri comunali, persone che si trovano

perché, additando tutto ciò che può essere in qualche modo sparso con il fango del ventilatore, travolgeremo i princìpi più importanti della nostra Costituzione: quel principio di sacra legalità

una sofferenza profonda perché quello che abbiamo fatto fino ad ora tocca solo in parte la questione. Anche se tutti gli interventi

quando capiremo tutti quanti che, al di là degli *slogan* che stanno uscendo in questi giorni («processiamo i colpevoli», «mandiamo tutti in galera», «la giustizia deve essere rapida, deve essere giusta»), la giustizia - attenzione, colleghi

la nostra professione, la nostra famiglia, le nostre relazioni personali rischiano di subire uno sfregio profondo a fronte di un semplice sospetto processuale; un sospetto processuale destinato a durare una vita intera. Colleghi, vi prego, qui siamo oltre il dibattito politico, stiamo trattando della vita delle persone, della carne e del sangue del Paese. Non dimentichiamoci mai di questo. Ricordiamoci che stiamo rappresentando gli italiani. Ricordiamoci di quella Costituzione che abbiamo visto criticare, qualche volta, alle inaugurazioni degli anni giudiziari in cui i magistrati sfilavano con il testo fondamentale in mano. Ecco, io credo che questi magistrati, io credo che questi avvocati, fortemente influenzati dal pregiudizio politico, quella Costituzione dovrebbero cominciare a leggerla. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Dovrebbero cominciare a capire che quello che c'è scritto non si applica a pezzatura di leopardo ma si applica sempre. Colleghi, voi sapete cosa vuol dire bloccare la prescrizione dopo il processo di primo grado? Questo è veramente il tema più significativo di questo sciagurato disegno di legge. Bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, significa che se il pubblico ministero appella voi, magari dichiarati innocenti in primo grado, continuate a rimanere appesi ad un filo, con la spada di FI-BP e della senatrice Bonino)*. Lo ripeto ancora una volta, colleghi, non sono solo parole. La giustizia è quella strana cosa che si capisce fino in fondo solo quando ti tocca personalmente. Il processo è quella strana cosa che viene avvertita come una bomba, un ordigno termonucleare, come ha detto la ministra Giulia Bongiorno senza essere però arrivata alle estreme conseguenze nel suo ragionamento, solamente quando esplode nel tuo salotto, non nel salotto degli altri. Amici, colleghi, Presidente, i tempi di un processo non sono indifferenti. Noi abbiamo assistito a delle barbarie giudiziarie, a persone che sono rimaste sotto processo per vent'anni per poi essere dichiarate innocenti nell'incuria, nel menefreghismo, nella totale indifferenza senatrice Bonino)*. Approvare questo provvedimento, questo testo significherebbe legittimare per sempre questa modalità. Non abbiamo bisogno di citare gli articoli della Costituzione che sono stati violati. Li conosciamo tutti e li abbiamo presenti, però vorrei ricordare a tutti noi, colleghi, credetemi senza alcuna assertività e senza alcuna arroganza, che noi tutti siamo qui come se avessimo moralmente e formalmente giurato sulla Costituzione che tante volte senatrice Biti)*. Vi prego, non mettiamoci anche stavolta in questa condizione dinnanzi al popolo italiano, l'unico con cui noi sentiamo di avere stipulato un contratto, perché a noi dei contratti di Governo non ce ne importa niente. Noi abbiamo

non deviazioni per ascoltare la voce del potere che ci tiene legati alle poltrone. Noi vogliamo fare bene, noi vogliamo fare in modo che i destinatari di queste leggi - cioè tutti noi - possano essere grati a questo Parlamento e orgogliosi di noi per aver fatto qualcosa di buono che impatta impatta immediatamente sulla vita dei cittadini. Purtroppo questo è esattamente il contrario di quello che stiamo facendo oggi. Noi abbiamo chiesto alla Camera dei deputati di poter intervenire su questo testo, di poter intervenire sulle parti peggiori di esso. Pensate, colleghi, che per la prima volta è capitata un'alchimia straordinaria, come ha ricordato, nella sua magistrale relazione di minoranza, il collega Caliendo: è successo che tutti, l'Accademia, gli avvocati, gli avvocati penalisti, i magistrati, tutti siano d'accordo nel dire che non si può modificare in questo modo il codice penale, il codice di procedura penale, l'assetto del processo, non si può condannare il cittadino italiano ad un ergastolo processuale infinito. Tutti lo dicono, anche i magistrati. Tutti dicono che l'effetto paradosso ottenuto da questo provvedimento, che vuole abbreviare i tempi della giustizia, è che in realtà li allunga drammaticamente, perché ciò che veramente allunga i tempi del processo - colleghi, guardiamoci negli occhi e diciamocelo chiaramente sono le lungaggini dei magistrati. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Di alcuni magistrati, non di tutti. Guardate la differenza tra le diverse procure e tra i diversi tribunali. Voi sapete - ce lo avete detto e ce lo siamo detti tra di noi - che il 70 dei procedimenti muore per prescrizione in fase di indagini preliminari. Che vuol dire, sono gli avvocati? Il ministro Bonafede curiosamente oggi non è presente. Il padre di questa legge abbia il coraggio di presentarsi davanti a questo Parlamento! chiedere, come immagino, la fiducia - atto di viltà - su questo provvedimento. Abbia il coraggio di presentarsi e di spiegare perché lui, avvocato, e il presidente Conte, avvocato, hanno detto che sono gli avvocati a rallentare i tempi del processo: amici, i tempi del processo in fase di indagine preliminare, quando ancora gli avvocati non sono stati messi in condizione di operare? *(Applausi del senatore Dal Mas).* Credetemi, non è una difesa di categoria, ma il ristabilire un principio di realtà.

I colleghi che mi hanno preceduto ne hanno citati alcuni. La senatrice Modena, giustamente, ha ricordato che qui si parla di provvedimento anticorruzione, ma noi dovremmo ricordare a tutti che i reati contro la pubblica amministrazione non sono solo la corruzione. La vogliamo smettere di parlare per etichette? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Vogliamo spiegare agli italiani che cosa stiamo facendo veramente? Alcuni aspetti di questo provvedimento risultano particolarmente inquietanti a chi, come noi, ha sempre combattuto per la libertà e per le garanzie. Noi non possiamo pensare che esista un soggetto legittimato dall'ordinamento giuridico a indurre qualcun altro a commettere un reato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Un agente sotto copertura? No, questo è un agente provocatore: è un soggetto che in un rapporto alla pari, faccia a faccia tra due persone, fa di tutto per indurre qualcun altro a commettere un reato, con la copertura dell'impunità. E questo quando lo stesso presidente Conte è venuto qui a dirci: mai e poi mai noi inseriremo nell'ordinamento l'agente provocatore.

avverto che, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale è stata richiesta da parte del prescritto numero di senatori la votazione a scrutinio segreto. Tale richiesta non può essere accolta in quanto l'articolo 93, comma 5, del Regolamento prescrive che il voto sulla questione pregiudiziale sia effettuato con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

che incide profondamente su tutti i diritti che il Regolamento menziona quali materia sulla quale si deve poter chiedere, con il prescritto numero dei senatori, il voto segreto. Il fatto che l'articolo 93, comma 5, del Regolamento

le leggi delega, vanno votate allo stesso modo, cioè con scrutinio simultaneo: vuol forse dire che se una legge viene fatta per delega e con quella legge si istituisce la pena di morte non ci può essere il voto segreto? È una cosa inaccettabile!

nell'approvazione del nuovo Regolamento è stato chiarito che sono cancellati tutti i precedenti. Poiché è nuovo il Regolamento, cambia la natura del Regolamento stesso, cambia il modo di lavorare e non può essere considerato valido alcun precedente.

credo che la Presidenza debba valutare molto più attentamente le questioni che sono state poste rispetto al voto segreto. Abbiamo già contestato le decisioni della Presidenza su situazioni, seppur diverse, che avevano però qualche analogia.

spaventata dai voti segreti su questo provvedimento, ha deciso di mettere la fiducia. Ha deciso di impedire un dibattito serio e approfondito su questioni delicate che riguardano i diritti dei cittadini. dai Gruppi PD e FI-BP)*. Noi concordiamo con la richiesta di riprendere l'esame di questa decisione, di permetterci, almeno su questo, il voto segreto, di interpretare correttamente il Regolamento e soprattutto di rispettare la libertà dei singoli Parlamentari, che ormai da questa maggioranza viene costantemente impedita per via delle paure delle loro divisioni.

Presidente, le chiederei la cortesia di sospendere la seduta, se possibile, e verificare, anche con il Presidente del Senato (senza nulla togliere naturalmente alla sua autorevolezza), se esistano le condizioni, in primo luogo, per la convocazione della Giunta per il Regolamento e, in secondo luogo, per rivedere la posizione che lei ha attualmente esposto. NENCINI

non volevo intervenire, ma non posso non farlo dopo le parole del Presidente del Gruppo Forza Italia che stimo e rispetto e ho sempre dimostrato di farlo. Credo non si possa mettere in dubbio

nelle condizioni di valutare le proposte che in questa sede sono state avanzate. Ricordo che le deliberazioni che si possono sottoporre al voto segreto devono riguardare oggetti che incidono su alcuni articoli della Costituzione. Qui stiamo parlando di una pregiudiziale e il voto non è nel merito del provvedimento,

questione del voto a scrutinio segreto e credo che si possa procedere in questa direzione.

Evidentemente ciascuno di noi ha opinioni diverse, ma è logico e ovvio, altrimenti voteremmo tutti allo stesso modo. Tuttavia, mi sembra che da parte del collega Malan sia venuta una richiesta molto seria, che a mio avviso è pregiudiziale rispetto al contenuto. Siamo in una fase nuova, di applicazione di un Regolamento nuovo; i precedenti sono stati, in qualche modo, annullati da un evento come il nuovo Regolamento; ci troviamo davanti a una fattispecie che presenta che presenta elementi di novità. Pertanto, con tutto il rispetto per la decisione insindacabile della Presidenza, che rispetto, anche se non la condivido,

il presidente Casini. È evidente, presidente Patuanelli, con il massimo rispetto anche per lei, che quando si parla di questioni pregiudiziali si tratta di pregiudizialità costituzionale, quindi ciò che viene chiamato in causa sono esattamente gli articoli della Costituzione contro cui contro cui questa norma, teoricamente, risulterebbe essere posta in essere. Ciò detto, ribadisco ancora una volta la nostra richiesta formale di convocazione della Giunta per il Regolamento, perché riteniamo che, a fronte di una questione che evoca e richiede la libertà di coscienza, la massima libertà di espressione dell'autonomia del parlamentare, non si possa che prevedere un'interpretazione del nuovo Regolamento del Senato nell'ottica della libertà e se questa interpretazione non va *de plano*, ma si ricollega a precedenti che sono decaduti

Presidente, ci troviamo ovviamente dinanzi a un fatto nuovo, come diceva il collega Casini, ossia l'applicazione di un nuovo Regolamento, per cui non possono essere invocati dei precedenti su questa fattispecie. ricordo un concetto che ha caratterizzato la nostra attività di parlamentari e anche la mia esperienza di Presidente del Senato e di Capogruppo. Il concetto era quello della valutazione della prevalenza.

Ora, non vi è dubbio che questa riforma tocchi un tema sensibile, che è quello della libertà del cittadino e dei diritti della persona, ed è un tema che, articolo per articolo, postula la possibilità di una richiesta di voto segreto. Se questo disegno di legge tocca, come tocca, nella sua effettività, questi princìpi, che sono quelli della inviolabilità o violabilità, secondo le sanzioni e le nuove norme precettive che si inseriscono, della libertà della persona, allora la prevalenza è quella del voto segreto.

un'eventuale pausa perché la stessa Presidenza possa consultarsi con il presidente Casellati sull'opportunità di convocare la Giunta per il Regolamento, che è un organo istituzionale in cui tutte le forze politiche sono rappresentate, sia una richiesta di buonsenso. È successo tante volte nella storia del nostro Parlamento, lei ricorderà che nella precedente legislatura si è riunita molte volte la Giunta per il Regolamento. Questo perché siamo dinanzi ad un fatto nuovo da un lato e, dall'altro lato, siamo dinanzi a un principio, che è quello della tutela della libertà della persona, che viene

La Presidenza ha preso una decisione. Come sanno anche i colleghi, la convocazione della Giunta per il Regolamento è esclusiva prerogativa del Presidente del Senato. Sospendo pertanto brevemente la seduta al fine di potermi confrontare con il Presidente per sapere se intenda o no convocare la Giunta per il Regolamento. *(La seduta, sospesa

La seduta è ripresa. Poiché è stata posta una questione interpretativa riferita all'articolo 93, comma 5, del Regolamento, così come modificato dalla novella del 20 dicembre 2017, ritengo opportuno, in assenza di precedenti e in ossequio al mio ruolo di garante della correttezza del dibattito parlamentare, convocare la Giunta per il Regolamento. A tal fine, poiché la Giunta A tal fine, poiché la Giunta era carente di due componenti, ho provveduto a integrarla nominando i senatori Stefano Patuanelli e Ugo Grassi,

intende che sia osservata questa pausa nel senso che era stata comunque determinata nella Conferenza dei Capigruppo, o se è disponibile a questa convocazione immediata della Giunta in Sala Pannini.

Adesso ci riuniamo immediatamente con la Giunta per il Regolamento per poter discutere sulla questione interpretativa posta.

a seguito delle richieste avanzate da alcuni Gruppi, ho convocato la Giunta per il Regolamento per esprimere un parere sull'ammissibilità del voto a scrutinio segreto sulla questione pregiudiziale. Nel precisare che, per ragioni di correttezza istituzionale, non ho partecipato alla votazione, comunico che tale richiesta di parere non è stata accolta dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento. Come ho anticipato nel corso del dibattito, il tema potrà essere nuovamente affrontato se vi saranno proposte di modifica del Regolamento al riguardo.

Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,

Regolamento del Senato, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento, ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento. La seduta è sospesa fino alle ore 16.

alle ore 16,06)*. Onorevoli colleghi, la Presidenza, ha esaminato l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 955. Tale proposta recepisce integralmente il testo della Commissione giustizia, pertanto la Presidenza ritiene ammissibile l'emendamento presentato dal Governo. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento e la la democrazia diretta**.* Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge

sostitutivo del disegno di legge al nostro esame, e trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia. La seduta è sospesa. La seduta è sospesa.

Per la discussione sulla fiducia, che si concluderà nella seduta odierna, sono state ripartite tre ore, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni di voto avranno invece luogo nella seduta di domani, con inizio alle ore 9,30.

del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 955. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

l'istituto della prescrizione e indicare nuove norme sulla tracciabilità dei finanziamenti al sistema dei partiti e dei movimenti politici.

non interviene, a nostro modo di vedere, nella giusta direzione, che deve essere una direzione garantista, una direzione garantista, possibilmente liberale, rispettosa dello stato di diritto e della nostra Costituzione. Ebbene, quest'oggi si sono votate due

acquisiscono l'ombrello delle protezioni costituzionali. Lo fate in modo maldestro, prevedendo un inasprimento delle pene accessorie a fronte di pene principali per reati di corruzione o reati attinenti alla pubblica amministrazione minimali: due anni e un giorno sono sufficienti per avere una condanna a una pena accessoria perpetua dell'interdizione dei pubblici uffici o un divieto perpetuo di contrarre con la pubblica amministrazione. Se questo lo vedo in relazione al traffico di influenze illecite, signor qualsiasi imprenditore si troverebbe davanti a una norma che prevede una pena accessoria per tutta la vita quando quella principale è una pena assolutamente modesta. Dov'è il principio di proporzionalità? *(Applausi Dov'è la Costituzione, signor ministro Bonafede? Prevedete poi la discrezionalità per i magistrati e questo è veramente un *unicum*. Il codice Rocco, in modo esplicito, stabilisce che la sospensione condizionale della pena principale comporta la sospensione della pena accessoria, voi invece introducete la possibilità per il giudice eventualmente di non sospendere la pena accessoria. Questa è veramente una previsione che va al di là del garantismo e anche della nostra immaginazione. Ad ogni modo, in tema di prescrizione le novità sono singolari, perché voi prescrivete la prescrizione

che nulla ha a che fare con l'azione penale. Se aveste voluto incidere sulla lunghezza dei processi, avreste dovuto incidere su ben altre norme, non sull'istituto della prescrizione che è un istituto a garanzia e a tutela dei cittadini, a garanzia e a tutela del diritto all'oblio, a garanzia e a tutela dello Stato quando non manifesta più alcuna utilità di carattere sociale nel perseguire un reato a distanza

dall'altro punto di vista, dall'altra parte della barricata, inteso come un meccanismo che, attraverso le impugnazioni,

sono convinto - che una parte di questa maggioranza, e non è un mistero quale sia (quella che esprime il Ministro della giustizia in questo momento in questo Paese) una visione che non è certo la nostra, che non è certo garantista, una visione massimalista, una visione giustizialista, una cultura del sospetto e nella cultura del sospetto voi pensate di costruire un sistema giusto, un processo giusto ed equo. Ebbene, state facendo esattamente il contrario. Pensate di intervenire sulla prescrizione pensando di intervenire nel processo penale rendendo il processo più agevole? No, di fatto - lo ha detto benissimo il nostro Capogruppo stamattina - voi mettete sulla testa dell'indiziato - imputato una spada di Damocle per tutta la vita e per di più lo fate anche rispetto a coloro che si ritengono persone offese

che sarà una causa di prescrizione della prescrizione perché il *dies ad quem* della sospensione coincide con l'irrevocabilità della pronuncia della sentenza di condanna o di proscioglimento

mi sarei aspettato che coloro i quali in ogni occasione dichiarano di essere i responsabili, i tenutari del cambiamento del Paese, intervenissero nel processo penale in modo importante e significativo, ma d'altronde abbiamo visto, e lo vedremo nella manovra di bilancio, che i primi tagli - circa 57 milioni - sono proprio destinati in gran parte alla riforma del processo penale. E se in effetti il tenore delle riforme che avete in mente è di questa portata, allora è da pregare Iddio che le riforme non le facciate, perché siamo seriamente preoccupati. L'articolo 530 del codice procedura penale dice che il giudice pronuncia la condanna quando vi è la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, noi abbiamo più di qualche ragionevole dubbio che questo sia un provvedimento illiberale, giustizialista e affetto da psicosi giustizialista.

Presidente, credo che il fatto che il Governo abbia posto la fiducia su questo provvedimento la dica lunga la dica lunga sulle difficoltà della maggioranza a stare insieme su questi temi. La dice lunga sul fatto che si pone oggi la fiducia perché non siete in grado di reggere i voti segreti che erano previsti, così com'è stato alla Camera: segno di una divisione della maggioranza seria, preoccupante. Guardate, questo è un dato politico: vuol dire che su questo provvedimento, materia del contratto di Governo,

sia alla Camera sia al Senato nella discussione di queste settimane abbiamo cercato di intervenire sul merito; non abbiamo mai preso posizioni Abbiamo cercato di spiegare le ragioni per cui questo provvedimento in molte sue parti è sbagliato, addirittura dannoso. Nelle scorse settimane noi abbiamo approvato in quest'Aula il cosiddetto decreto sicurezza, nome importante che caratterizzava il provvedimento. Noi abbiamo spiegato che per noi quella era una legge manifesto, una legge bandiera, la legge bandiera della Lega che doveva dimostrare al proprio elettorato l'attenzione a un tema che è stato molto utilizzato in campagna elettorale. Ma abbiamo anche detto che quello non è un provvedimento che darà o garantirà

che migliorino il controllo delle nostre città o che affronti meglio il tema di come tutelare i nostri cittadini per dare loro ancora più sicurezza. Si tratta di una legge che serviva e serve a dare alcune suggestioni, a parlare alla pancia del Paese; una legge che in realtà, ad oggi, ha prodotto solo quei danni che purtroppo avevamo previsto avrebbe fatto. Ci avevate detto che non sarebbe successo a invece ci sono in strada famiglie, persone che erano ospiti nei centri e che sono state messe in strada,

Oggi discutiamo e domani voteremo con la fiducia un provvedimento che nella sua filosofia non è tanto diverso. Anche questo è un disegno di legge con un nome impegnativo: «anticorruzione». In realtà però è un'altro provvedimento che serve a una parte di questa maggioranza, al MoVimento 5 Stelle, per parlare agli elettori, non per risolvere e affrontare i problemi dei cittadini.

combattere la corruzione per noi è una priorità, ma se confrontiamo le leggi che abbiamo fatto nella scorsa legislatura con questa leggina, allora

la possibilità di intervenire sui capitolati d'appalto prima che avvengano le gare? I poteri all'ANAC chi li ha dati?

troppo lievi? E, ancora, chi ha deciso che ai reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio debbano essere estese le misure che riguardano la confisca dei patrimoni? Tutto questo è stato fatto. Prima di dire che questa è la prima, la più importante e la migliore legge anticorruzione fatta in questo Paese, ricordiamoci queste cose, perché con questo provvedimento, anziché

Che senso ha spiegare che i corrotti, una volta condannati, devono essere esclusi dalla possibilità delle pene alternative? Che senso hanno Che senso hanno gli agenti provocatori, perché di questo stiamo parlando? O l'uso indiscriminato dei *trojan*? Lo Stato non è più forte se baratta libertà in nome della sicurezza, come abbiamo detto nelle scorse settimane, né è più forte se riduce libertà, garanzie e diritti per dare l'idea di contrastare un reato, certo odioso, come la corruzione. Uno Stato così non è più forte, semmai è più autoritario e meno liberale. Che idea sta sotto la scelta di bloccare le attività di un'azienda con la pubblica amministrazione, appena si prefigura - solo si prefigura una notizia di reato? È un'idea, la vostra, che risponde alla rabbia legittima di tante persone di fronte alla corruzione, ma la cavalca e non la risolve. Ricordatevi che aumentare la cultura del sospetto è il contrario di ciò che deve fare uno Stato di diritto. Che senso ha intervenire così sulla prescrizione? Si è appena fatta una riforma. Perché, se non per strumentalità politica, non aspettiamo di vedere gli esiti di quella riforma? Tanto più che poi dite che cambiate la prescrizione, però la fate entrare in vigore soltanto nel 2020, perché entro tale anno si pensa che faremo una riforma della giustizia che risolverà in pieno tutti i problemi

È un imbroglio questa legge, in cui il punto non è difendere la legalità, ma il messaggio che volete dare agli italiani: voi odiate i corrotti e noi, in nome di questo giusto sentimento, ci sentiamo legittimati a stravolgere lo Stato di diritto, a incidere sui sistemi delle garanzie per i cittadini, a a mostrare il volto di uno Stato che non persegue solo i colpevoli, ma che sospetta di tutti. Mi rivolgo a tutto il Governo: basta sacrificare i principi di uno Stato democratico e liberale, basta! Non potete farlo per soddisfare le vostre esigenze di partito, per soddisfare la vostra propaganda.

usciti dopo interminabili e infernali anni dalla gabbia giudiziaria in modo assolutamente innocente (e sottolineo, in modo assolutamente innocente), saremmo ancora prigionieri

e, come è capitato a me e a molti altri, saremmo, nell'attesa, oggetto di una ferocia mediatica, di un livore moralistico spregiudicato; saremmo oggetto di un «Vaffa penoso quanto umiliante, che la sua parte politica conosce bene, per averlo praticato con una intensità bugiarda e vanitosa, ma doloroso, ingenerosamente doloroso per chi lo subiva. Colleghi della maggioranza, questa giustizia è forse la vostra giustizia, ma non quella che racconta la nostra Costituzione. Il drammatico e aberrante emendamento che avete presentato è solo che avete presentato è solo una irresponsabile proposta di riforma, inutile quanto dannosa, inefficace quanto improduttiva ai fini del superamento della lentezza processuale. Non voglio essere irriverente, signor Ministro, ma le hanno mai parlato di ragionevole durata del processo? Le hanno mai detto che esistono diritti di imputati che lei considera eternamente colpevoli e non presuntivamente innocenti? Siamo passati con lei dal populismo giudiziario all'intimidazione Ci sarà una ragione per la quale - se l'è chiesto? - magistrati e penalisti sono concordi nel ritenere come la sua riforma sia fuori luogo, fuori misura, fuori tempo. Insomma, sia fuori.

per tutta la vita e sottolineo per tutta la vita. Sto guardando in questo momento tra i banchi del Governo per vedere se c'è il ministro Bongiorno, ma non c'è e la cosa mi dispiace. Anche se non c'è, a lei vorrei chiedere: ma avete disinnescato la bomba atomica messa nel processo? Fu Fu questo il linguaggio da lei usato per dimostrare la sua contrarietà nei confronti dell'emendamento Bonafede. Signor ministro Bongiorno, ha fatto marcia indietro? Cosa è cambiato? Ce lo spieghi. Il contratto di Governo supera anche il diritto, anche quello universale? Vuol dire che la Lega voterà a favore? Certo che lo farà, rendendosi corresponsabile di un delitto contro la Costituzione. Certo, avete messo la fiducia e questo racconta tutto. Avrei sperato che ciò non fosse successo e spero ancora - è un lumicino di speranza, visto come si sono messe le cose - che quanti in questa Aula credono ancora in ciò in cui hanno sempre creduto, ai valori primari della Costituzione, si ribellino e votino secondo coscienza dicendo no a una riforma che dà i brividi. Ma la vedo una cosa impossibile

e a essa non si sarebbe dovuto rinunciare. Così facendo, avremo sotto ricatto processuale permanente un cittadino a tempo indeterminato. E così purtroppo sarà. Visto che questa legge passerà - perché cari colleghi, sicuramente passerà - resta una sola speranza: mi auguro che il Capo dello Stato e la Corte costituzionale intervengano e che non lascino correre facendo finta di niente. Se così non fosse, ma non credo conoscendo la saggezza del presidente Mattarella e il rigore della Corte, non avremo altra possibilità se non quella di trovare un rifugio dove ancora le libertà siano i connotati fondamentali che presiedono alla vita civile. Ministro Bonafede, concludo ricordando a me stessa e a tutta questa

Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, da decenni il Paese attendeva un provvedimento come questo e finalmente adesso è qui, a ulteriore riprova del nostro impegno sul fronte dell'onestà e della legalità. Il disegno di legge n. 955 reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici. Come consuetudine, a ogni importante testo di legge viene attribuito un nome colloquiale che ne racchiude l'essenza e la comunica in modo semplice ai cittadini. In questo caso il soprannome spazza corrotti rende perfettamente l'idea dell'obiettivo che questo provvedimento si prefigge: la necessità di fare pulizia e di eliminare la corruzione dalle strutture amministrative che costituiscono la spina dorsale del nostro sistema economico. Sì, perché la corruzione perpetrata all'interno della pubblica amministrazione è un virus malefico che avvelena e indebolisce l'economia del nostro Paese. Molteplici studi, tra cui quello effettuato da Unimpresa, hanno dimostrato che il peggioramento di un punto dell'indice di percezione della corruzione determina una riduzione annua del prodotto interno lordo pari allo 0,39 Ciò significa che nell'ultimo decennio la corruzione è costata all'Italia 100 miliardi di euro. E questo è solo il primo punto della lunga lista di danni economici causati dalla corruzione al nostro Paese. La corruzione, infatti, allontana gli investimenti stranieri, in particolar modo quelli sani, lasciando la strada aperta agli imprenditori imprenditori senza scrupoli e avvezzi all'utilizzo delle mazzette; rallenta la crescita delle imprese, perché le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25 per cento in meno rispetto a quelle operanti in un contesto di legalità; distoglie gli investimenti nei confronti dell'innovazione e della ricerca, togliendo competitività alle imprese. Infine, allungando i tempi della burocrazia, danneggia l'efficienza del nostro sistema produttivo. La corruzione non si limita solo a ledere il nostro sistema economico; essa ha un impatto rilevante anche sul tessuto sociale. Questo è forse un male ancora peggiore perché compromette la fiducia dei cittadini nello Stato, che non è più visto come il garante imparziale dei diritti di tutti, ma come un coacervo di poteri in vendita al miglior offerente. risorse da spendere in tangenti ha la possibilità di influire sulle decisioni dei funzionari pubblici, gli altri restano fuori. E non si parla soltanto di episodi sporadici ed eclatanti, non si parla dell'orrore degli appalti truccati che producono scuole che crollano sulla testa dei nostri figli o di strade che si sgretolano sotto i nostri si parla anche della miriade di piccoli episodi che punteggiano la vita quotidiana di milioni di cittadini, che ormai trovano normale rivolgersi ai potenti di turno per trovare un lavoro o ricevere una prestazione sanitaria in tempi decenti. Ma tutto questo però non è affatto normale, non può e non deve essere

affinché tutto ciò avvenga è portare alla luce i fatti di corruzione. A questo proposito è fondamentale l'estensione della figura dell'agente sotto copertura, già utilizzato per la lotta al terrorismo, alla droga e alla criminalità organizzata, utilizzandolo anche in materia di corruzione nella pubblica amministrazione. Tale soggetto avrà la possibilità di osservare direttamente le trattative tra corrotto e corruttore e fornirà la testimonianza di azioni che altrimenti non avrebbero la possibilità di venire a galla. Appartenente alle Forze dell'ordine, l'infiltrato potrà vestire i panni di un impiegato pubblico o privato, che osserva e riferisce tutto agli inquirenti, raccogliendo le prove necessarie ad incastrare i corrotti. Pertanto, attraverso l'articolo 6 si estende la disciplina delle operazioni sotto copertura al contrasto della corruzione, proprio perché, al pari dei reati prima indicati, la stessa si nutre di omertà. potrà essere efficacemente combattuta. Con la modifica introdotta dall'articolo 6 nessuno sarà più sicuro di farla franca. Nello stesso alveo concettuale debutta la figura del pentito della corruzione. Infatti, con l'articolo 1, comma 6, lettera *s)*, viene introdotta una nuova ipotesi di non punibilità. Con l'inserimento dell'articolo 323-*ter* non sarà punito chi, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato ed individuare eventuali altri responsabili. Occorrerà però inoltre, per beneficiare della non punibilità, che il pentito della corruzione restituisca l'utilità percepita o una somma di denaro equivalente. Un altro fondamentale strumento per la lotta alla corruzione è anche l'esclusione dei corrotti dalla pubblica amministrazione. Chi verrà condannato dovrà essere escluso e non potrà quindi più partecipare ad appalti pubblici. Ci sono quindi una serie di strumenti che permetteranno l'inasprimento delle pene e quindi il cosiddetto spazza corrotti viene inteso non come un semplice disegno di legge, ma come una riforma strutturale in grado di restituire competitività al Paese e di operare il e di operare il cambio culturale necessario a rimettere l'Italia sui giusti binari della legalità. Il cambio di rotta e di mentalità è quello che gli italiani ci hanno chiesto e quello che essi si aspettano dal Governo del cambiamento. Non è più tempo di fare i furbi. Cambiamo questo distorto concetto di furbizia e cominciamo a chiamare i corrotti e corruttori con il vero nome: ladri.

di questi principi perché in essi crediamo fortemente. Tali principi sono legati a battaglie di giustizia e di libertà che abbiamo combattuto da tempi non sospetti. Qui si vuole cambiare un principio, che non è che sia nato ieri, che sia piovuto dal cielo o che sia saltato fuori come Minerva dalla testa di Giove;

per tutti i reati, ad esclusione dell'omicidio. I reati nell'antica Grecia si prescrivevano in cinque anni. Questo è un elemento che dovrebbe far comprendere a quest'Aula l'importanza di un istituto che non è stato inserito all'interno del nostro ordinamento in maniera casuale. Le cause di estinzione del reato, dalla morte del reo alla remissione della querela addirittura all'applicazione di altre norme, come ad esempio l'amnistia propria, sono cause di estinzione del reato e della pena.

culturale perché ho l'impressione che lei, signor Ministro, abbia origini culturali di stampo giansenista: come lei ricorderà benissimo, Giansenio pensava che l'uomo fosse nato corrotto e cattivo e che in qualche modo

Un personaggio, che è forse l'ispiratore di questa manovra, Piercamillo Davigo, ripeteva che non ci sono innocenti, non esistono:

genitori, gli affetti più cari e c'è un fine pena mai, in un tempo immobile, in attesa di non sappiamo cosa, anche per gli innocenti, nel momento in cui il pubblico ministro Ministro, quando lei all'inizio ha detto che ci sarebbe stata questa riforma, pensavamo che fosse una *boutade*, qualcosa tipo le scie chimiche che ci avete ricordato all'inizio, durante la campagna elettorale. Secondo me, signor Ministro, lei vive in un mondo popolato da colpevoli. Noi invece pensiamo che il nostro mondo sia popolato solamente da esseri umani che necessitano, non solo di comprensione, ma di rispetto, soprattutto del prossimo. Non possiamo seguire questa deriva. Sarebbe già stata sufficiente la riforma Orlando, signor Ministro: diciotto mesi di sospensione dopo il primo grado e altri diciotto dopo la sentenza di appello. Ripeto, sarebbe stata sufficiente.

che magari hanno qualche problema oggi; riguarderà tutti, riguarderà i familiari e tutti coloro che vengono coinvolti, magari loro malgrado, in un procedimento penale, che non vedrà mai la fine. Sono

È esattamente il contrario. L'unico pungolo che abbiamo, l'unico strumento che esiste per accelerare i tempi di definizione di un procedimento è quello di prevedere per ogni *step* la prescrizione, tant'è che è un istituto a salvaguardia di un altro principio, quello della ragionevole durata del processo, previsto all'articolo 111 della Costituzione. Mi permetto di dire che questo articolo è stato inserito per contemperarne un altro,

finisce per estinguersi, non per responsabilità degli avvocati, degli imputati e degli indagati, ma perché le procure della Repubblica e gli uffici del GIP non riescono ad arrivare al termine. Lei, signor Ministro, ha ha detto che è finita l'era dei furbi e degli azzeccagarbugli e questa frase, signor Ministro, non le fa onore. Io ho indossato, come tanti colleghi, quella toga quella toga che ha portato alla difesa dei principi e dei valori costituzionali, non solamente degli imputati, ma in tantissimi casi anche delle persone offese, di chi chiede giustizia in Italia. Questo è un aspetto che dobbiamo anche prendere in considerazione, cioè il dileggio che si è dato alla nostra categoria. Dobbiamo riconoscere un miracolo: il miracolo di "San Bonafede". Signor Ministro, con quest'operazione lei a mettere d'accordo tutti coloro che erano su posizioni diametralmente opposte: avvocati, magistrati, coloro che sono operatori nell'ambito del diritto nelle università. se vogliamo varare una vera riforma organica, incominciamo col dire che dopo che si viene assolti in primo grado non c'è più la possibilità di fare appello. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Diciamo ancora che quando si entra nelle aule giudiziarie non si deve dare del lei, come fanno gli avvocati, al pubblico ministero e al giudice,

un problema di poco conto. L'eliminazione della prescrizione è un problema che riguarderà ognuno di noi, che deve riguardare ognuno di noi, che deve portare le nostre intelligenze a comprendere l'importanza di un voto negativo su quello che state facendo, perché così veramente forse aveva ragione la sua collega Bongiorno - avete innescato un ordigno nucleare all'interno del processo penale. Sta a voi in questo momento disinnescarlo. Noi abbiamo fatto il possibile in quest'Aula con gli interventi facciamolo non solamente per una parte politica, ma in difesa nell'Italia, dei valori che hanno sorretto il nostro ordinamento e soprattutto di quello che dicevo prima: la nostra Italia, culla del diritto. Non stupriamola così, signor Ministro.

è particolarmente vera per il particolare di cui desidero parlare nel caso del disegno di legge che stiamo discutendo e lo è ancor di più in relazione all'articolo 6, all'articolo 6, che estende la speciale causa di non punibilità prevista per gli agenti sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione, una misura che in linea di principio non risulta a prima lettura irragionevole, ispirata ad irrobustire le azioni di prevenzione e contrasto a questo tipo di reati.

Mi riferisco, in particolare, alla saldatura tra l'estensione dell'impiego di agenti infiltrati ai delitti di corruzione e l'applicazione della causa di non punibilità alle attività prodromiche strumentali. Non è una questione di lana caprina, signor Ministro. Per ventidue anni io ho servito la mia città. Ho fatto la consigliera comunale e ho conosciuto a fondo gli uffici di una grande città e di un grande Comune quale quello di Roma e questa non è una questione da prendere sottobanco. C'è una distinzione importante da fare: bisogna fare molta attenzione, cari colleghi, quando si decide di prevenire e reprimere reati facendo ricorso all'opera di agenti infiltrati. È necessario, infatti, tenere ben distinta la figura dell'agente sotto copertura, che interviene quando la condotta criminosa è già definita ed è già in atto. Condotta, mi insegnava il mio grande maestro di vita e di libertà, Franco Cordero, vuol dire fatto. Ce l'abbiamo, nella fattispecie che specifica il principio del *ne bis in idem* dell'articolo 90 del codice di procedura penale. ma vuol dire che quel fatto è già *in itinere*, che quella condotta di reato già esiste. Mentre è molto diversa la figura dell'agente provocatore,

Attenzione su questo. La figura dell'agente provocatore contrasta profondamente con l'elementare principio dello Stato di diritto. Penso alla responsabilità penale, che è personale. Lo sappiamo a memoria, tutti noi che abbiamo studiato diritto penale e io che l'ho insegnato per tanti anni. Parlo la responsabilità penale è personale. Ma, più in generale, penso anche al contrasto con il ruolo che uno Stato fiducioso delle proprie capacità deve assumere nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Uno Stato serio, signor Ministro, previene, reprime, protegge le vittime del reato e costruisce le condizioni per il reinserimento del reo; non induce i privati cittadini a commettere dei reati. Riflettete su questo. Riflettete su questa situazione. Pensate alle conseguenze aberranti, specie laddove il confine tra lecito e illecito sia sia di difficile individuazione, sia difficile da cogliere o laddove più alto sia il rischio di delazioni. Ancora, signor Ministro, io la invito a ragionare sulle conseguenze di una simile previsione nelle amministrazioni collocate in territori difficili e particolari. Penso a tanti sindaci e a tanti piccoli Comuni. Ma davvero, signor Ministro, lei cosa vuole? Vuole trasformare gli uffici delle pubbliche amministrazioni in un luogo di spioni, di delatori, di gente che si invidia e si mette l'uno contro l'altro, che instilla chissà quale dubbio, magari solo per invidia di un collega? Attenzione, perché questo è quello che voi perpetrate in ogni atto che fate, sottacendolo, ma manifestandolo poi concretamente: fomentare quell'odio, quel rancore sociale e quell'invidia solo magari perché una una persona è arrivata dove un'altra non può o non è riuscita ad arrivare. Sarebbe stato meglio confrontarsi. Guardi, signor Ministro,

questa roba in Commissione c'è stata un pomeriggio e una notte. Vedo il collega Caliendo, la collega Modena, il mio capogruppo Cucca; non c'è stata discussione, non c'è stato approfondimento. E ora la fiducia cala come una scure; signor Ministro, questo non va bene. Sarebbe stato meglio confrontarsi, non porre la fiducia. Ma voi l'avete posta per paura; per paura della tenuta della vostra maggioranza. Non a caso i banchi della Lega sono quasi tutti vuoti e ci siete solo voi, che caparbiamente volete questo testo per fare l'ennesimo lavaggio del cervello, utilizzando un lessico che fa sdegno a chi ha insegnato per tanti anni in un'università, come me: Ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa spazzate? Signor Ministro, lei, che ha rappresentato l'avvocatura in un foro importante come quello di Firenze, dove la lingua italiana è nata e dove ne abbiamo «lavato i panni in Arno» la smetta di usare questi termini offensivi per il Paese dove è nato il diritto. Concludo, signor Presidente, dicendo che sarebbe stato meglio, senza pregiudicare l'estensione dell'uso di agenti sotto copertura anche nel contrasto ai delitti di corruzione, eliminare le attività prodromiche e strumentali alla commissione di reati dalle condotte scriminate, per consentire una migliore delimitazione della fattispecie, tenendo in piedi la tipizzazione già esistente. L'hanno citata i colleghi che hanno parlato prima di me: l'aveva già sufficientemente bene la riforma fatta dal ministro Orlando. Sarebbe stato un intervento minimo, ragionevole, che potevamo discutere e accogliere con un emendamento, da cui avrebbero potuto avere beneficio due importanti principi: sia lo Stato di diritto, che per noi conta molto (per voi forse di meno) nell'equilibrio tra garanzia e legalità sia la tutela dei diritti fondamentali. Il voto di fiducia non consente emendamenti e blinda questo testo: un testo pessimo e anticostituzionale.

Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, era il 17 febbraio 1992 quando veniva arrestato Mario Chiesa; da lì iniziò Mani pulite, cioè quella serie di inchieste che portò alla luce un sistema fraudolento che coinvolgeva politica e imprenditoria. Da quel momento l'Italia capì di avere un vero e proprio problema sociale: la corruzione. Oggi, a distanza di ventisei anni, è a dir poco drammatico realizzare che la situazione è cambiata nei minimi termini. Oggi, a distanza di ventisei anni, con la sua incidenza sul PIL nazionale di circa 10 miliardi di euro l'anno, la corruzione produce ancora più danno economico di allora. E, se studiamo il fenomeno corruzione in Italia, data la sua stretta connessione con il mondo politico, non fosse altro perché è la politica a dare i mezzi per combattere il fenomeno e magari a reprimerlo,

Oggi arriva la risposta. Oggi noi, con questa legge, dimostriamo cosa deve fare una forza di maggioranza, cioè il contrario di quello che ha fatto, o meglio che non ha fatto, la politica degli ultimi vent'anni, quella che immediatamente dopo Mani pulite, immediatamente dopo le stragi di mafia, invece di dotarsi di un sistema efficace di leggi per debellare mafia e corruzione, non ha fatto altro che portarci in una condizione peggiore rispetto a quella di quegli anni Novanta. Lo testimoniano le notizie di cronaca e i dati economici di un Paese che vede, tra gli ostacoli alla crescita, proprio quello il malaffare. A nulla sono valse le indicazioni del Consiglio d'Europa e i richiami dell'OCSE. È strano che, quando si tratta di applicare le politiche di *austerity*, «ce lo chiede l'Europa»; quando invece si tratta di fare una legge seria contro la corruzione, non ce lo chiede l'Europa. Eppure ce lo chiede da tempo. È sotto gli occhi di tutti che qualcosa non funziona: bisogna intervenire subito. Il sistema di corruzione vigente nel nostro Paese si fonda su tre pilastri, ovvero: poche possibilità che questo tipo di reato venga scoperto;

grazie all'uso di agenti infiltrati, collaboratori, intercettazioni e custodia cautelare in carcere. Il blocco della prescrizione dopo il primo grado darà la certezza di giungere a una sentenza definitiva, visto che nessuno avrà più interesse a rinviare alle calende greche il proprio processo, non potendo più contare proprio sulla prescrizione. Le pene più alte, infine, renderanno reale l'eventualità di non restare impuniti. Con il disegno di legge al nostro esame interveniamo anche sulla trasparenza dei finanziamenti ai partiti, in modo che i cittadini sappiano chi finanzia quale partito. Oggi si mette la parola fine a quella che è diventata ormai una prassi di degenerazione spirituale e morale, di vera depravazione, che porta effetti devastanti sull'economia del Paese, non soltanto per ciò che riguarda il PIL, ma anche sul costo degli appalti e sul *trend* degli investimenti esteri, che da sempre Si tratta di effetti, che si riversano inesorabilmente su tutti gli altri comparti, a iniziare dal lavoro,

la Basilicata è la mia terra. Oggi, con una Giunta regionale indagata per abuso d'ufficio, con un presidente sospeso, prima agli arresti domiciliari, oggi sottoposto a divieto di dimora nel capoluogo di Potenza, è una Regione tra le più corrotte in Europa. Questo è il responso severo dato dal Quality of government institute della facoltà di Scienze politiche dell'università svedese di Göteborg, che periodicamente effettua rilevazioni sulla qualità della pubblica amministrazione europea, analizzandola sotto tre aspetti: qualità, imparzialità e (indovinate un po'?) corruzione. Non a caso, signor Presidente, in Basilicata si muore di tutto, dall'inquinamento alla disoccupazione, dai cattivi servizi alla mancanza di infrastrutture. Il risultato è che la mia Regione, in dieci anni, ha perso il 10 per cento della popolazione, in maggioranza giovani. Ecco cosa produce la corruzione.

ricordando a tutti i colleghi dell'Assemblea, indipendentemente dal colore politico, che senza legalità non ci potrà mai essere sviluppo nei territori.

il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati (…)» è «di condannare i deboli innocenti»; «ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico». Ebbene, il disegno di legge in esame contraddice tutti e tre questi principi FI-BP)*perché la pena avviene lontanissima dalla commissione del delitto, con processi infiniti, i deboli innocenti vengono afflitti tanto e più dei robusti scellerati, perché un innocente deve aspettare decenni per avere la giusta sentenza, mentre al colpevole conviene benissimo aspettare: meglio aspettare, anche perché, giustamente, prima di una condanna definitiva non si può finire in carcere se non per le misure cautelari, che dovrebbero essere limitate il più possibile. Pertanto qui si tutelano i colpevoli e si condannano gli innocenti.

Poi, dopo vent'anni, si scopre che quella persona era innocente, ma intanto la sua vita è distrutta e i suoi dipendenti a casa anche loro, perché è giusto, non è vero? È giusto distruggere le aziende sulla base del sospetto, perché i processi devono durare cinquant'anni, perché volete

e sono state scritte più di duecentocinquant'anni fa: facciamo un balzo secolare all'indietro con questo provvedimento. Il senatore Aimi ha ricordato che anche nell'antica Grecia si prescrivevano i reati in cinque anni; ci possono essere esempi anche molto celebri, ma restando nell'antica Grecia, come disse Pericle, noi non abbiamo paura della discussione perché non riteniamo che la discussione sia un ostacolo alle giuste decisioni; riteniamo piuttosto che sia il modo giusto per prenderle. Quello che oggi è avvenuto è che avete troncato la discussione; avete impedito a quest'Assemblea di intervenire; il 92 per cento dei senatori non ha potuto fare nulla su questo provvedimento perché non fa parte della Commissione giustizia.

anche l'agente provocatore: una mostruosità. Lo Stato, se ha ragion d'essere, se è al servizio dei cittadini - come noi di Forza Italia abbiamo sempre creduto

Chi lo fa in queste vesti può compiere reati e non è punibile. Leggete l'articolo: non è punibile chi compie una serie di reati allo scopo di indurre altri a farne perché lo Stato, che si mette al posto di Dio, vuole punire, vuole giudicare il suo cuore, e non le sue azioni! dal Gruppo M5S).* Oltre ai principi, dei quali evidentemente a molti non interessa nulla, c'è anche l'economia: non solo i magistrati, gli avvocati, i costituzionalisti hanno espresso giudizi estremamente negativi su questo disegno di legge, ma anche le associazioni imprenditoriali,

ti può capitare una vicenda giudiziaria, può capitare a un tuo dirigente, e non puoi fare nulla perché per decenni il processo andrà avanti, l'assoluzione arriverà decisamente morta e pertanto è meglio andare in altri Paesi. Aggiungo un elemento: la perseguibilità d'ufficio della corruzione fra privati. In altre parole, sarà un magistrato a stabilire se un dipendente è stato fedele alla sua azienda e non il titolare della stessa azienda. FI-BP)*. Un imprenditore potrà vedere condannato uno dei suoi dirigenti o un suo impiegato, pur ritenendolo lui preziosissimo, perché a giudizio del signor magistrato non è stato sufficientemente ligio. Questa, oltre ai processi, è una bomba sotto le aziende. Ministro, legga quello che c'è scritto nel provvedimento. Apprezzo che lei segua - cosa che molti suoi colleghi non fanno anche quando vengono qui - però deve leggere quello che c'è scritto.

perché quando un magistrato fa un danno, quando distrugge la vita di un cittadino innocente, a poco serve che quello che giudica la causa accanto sia equanime e faccia le cose come si deve. La prescrizione serve anche a questo.

Un'Italia dove chiunque può essere messo in carcere e soprattutto sottoposto a processi infiniti, un'azienda deve rendere conto ad altri, naturalmente deve rendere conto alla legge ma deve sperare anche che nessun magistrato entri nei suoi meccanismi per stabilire se il tale dirigente ha fatto bene a rifornirsi da questo o da quest'altro fornitore, altrimenti è infedele,

inoltre, che se voi votaste contro questo provvedimento andreste incontro a delle conseguenze tutte politiche (spero solo politiche), per esempio quella di non essere ricandidati. Io però preferisco essere l'ultimo dei cittadini in un Paese dove vige lo Stato di diritto e dove la libertà dei cittadini è un valore supremo che senatore in un Paese dove lo Stato di diritto non c'è più.

questa mattina, intervenendo in sede di votazione della questione pregiudiziale posta dai Gruppi Forza Italia e PD, ho annunciato il voto di astensione di Fratelli d'Italia, auspicando che il Governo e la maggioranza accogliessero il nostro invito a confrontarci nel merito; pochi minuti dopo il Governo ha posto la fiducia, dimostrando di non avere alcun interesse al confronto nel merito. Questa è la risposta ad un atteggiamento costruttivo

per la lotta alla corruzione. Ricordo che Fratelli d'Italia è in prima linea nella lotta contro la corruzione che avvelena l'economia, la libera concorrenza e il Paese intero. Esso contiene, inoltre, alcune misure

la maggioranza e il Governo sono rimasti sordi e si sono rifiutati, prima in Commissione e poi in Aula, di affrontare i nostri emendamenti, tutti migliorativi del disegno sono rifiutati di affrontare il grido di allarme che noi, come altri Gruppi, abbiamo lanciato su questa riforma, anzi su questa controriforma in materia di prescrizione. Una riforma pericolosa, signor Ministro, una riforma che viola elementari principi acquisiti da secoli nella nostra civiltà giuridica, una riforma che va contro il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, che va contro l'articolo 6 della Convenzione europea per la che sancisce il diritto del cittadino ad avere un processo rapido ed efficace, il diritto del colpevole come dell'innocente, il diritto dell'imputato a non essere sottoposto a un procedimento penale infinito. Avremo il paradosso, signor Ministro, che tra poche ore lo Stato italiano avrà, da un lato, una norma che consentirà di rimandare all'infinito di rimandare all'infinito i procedimenti penali e, dall'altro, una legge che sanziona lo Stato se quel processo durerà più di sei anni (la cosiddetta legge Pinto): un atteggiamento puramente schizofrenico che farà storcere il naso a tutti i giuristi del del mondo. Quindi si tratta di una riforma che viola gli elementari principi della nostra civiltà giuridica. In cambio di che cosa? Fosse almeno utile, signor Ministro. Ma voi sapete benissimo che la riforma è anche inutile: cento dei procedimenti penali si estingue in istruttoria - lo ha detto il suo Ministero - e su questi la legge non interviene. Le dirò di più: secondo i dati Eurispes pubblicati qualche giorno fa dal «Corriere della Sera» un altro buon 10 per cento si prescrive entro la sentenza di primo grado (arriviamo all'80 per cento), e su questi il suo provvedimento non interviene.

a rivedere il suo giudizio assolutamente ingeneroso nei confronti dei difensori che svolgono un ruolo costituzionalmente garantito nell'interesse della libertà dei cittadini. Non c'è processo, non c'è civiltà giuridica senza la difesa, a meno che lei non pensi che sia sufficiente l'accusa per poter

Su cento rinvii nel processo penale solo il 3,6 per per ragioni legate al difensore e all'imputato, e in quel caso c'è anche la sospensione della prescrizione, mentre in tutti gli altri casi i rinvii sono dovuti ad errori del pubblico ministero che non cita i testi, a impedimento del giudice mille altri motivi che non hanno nulla a che vedere con la difesa, signor Ministro. Non sono azzeccagarbugli gli avvocati, bensì attori fondamentali del processo penale che meritano rispetto soprattutto da chi amministra la giustizia

risolto allungando all'infinito il termine della prescrizione, ma intervenendo sui problemi che hanno alcuni determinati - e ben - individuati sulla base delle vostre tabelle - uffici giudiziari, con più assunzioni, con più giudici, magari sottraendo qualche decina o qualche centinaio di giudici da compiti non legati alla loro funzione, dai Ministeri e da tutt'altre faccende che non hanno niente a che vedere

depenalizzazione; aumentando i procedimenti puniti a querela. Faccio solo un esempio: com'è possibile che oggi ancora in Italia le molestie telefoniche debbano essere perseguite d'ufficio? Questa è una cosa che sinceramente mi sfugge. E non è vero, signor Ministro, che allungare all'infinito, anzi eliminare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, serva a punire i reati contro la pubblica amministrazione. Non è vero e ce lo dicono le vostre tabelle: appena l'1 per cento dei reati contro la pubblica amministrazione finiscono prescritti nel corso del giudizio. E non potrebbe essere diversamente; lo dico anche al collega del MoVimento 5 Stelle che è intervenuto poco fa. Ma vi rendete conto che, anche per effetto della riforma Orlando, per prescrivere il peculato ci vogliono sedici

Se la giustizia non riesce a dare una risposta in una vita intera, voi pensate di risolvere il problema eliminando la prescrizione, che è un elementare principio di diritto e di giustizia che esiste dall'antica Grecia, come sottolineava giustamente il collega Aimi. Agli amici della Lega, stranamente silenti in questo dibattito, vorrei fare una domanda sola: com'è possibile che la bomba nucleare in una notte si sia trasformata in un petardo di carnevale? Com'è possibile che la bomba nucleare che doveva deflagrare all'interno del processo penale, secondo le esatte parole del ministro Bongiorno, in una notte si sia trasformata in un petardo? Anzi, nemmeno più in un petardo, visto il vostro silenzio, ma in un *flatus vocis* e nulla più. Ecco su questo, caro Ministro, non ci stiamo,

dell'agente infiltrato bastava fare una semplicissima norma dicendo che ciò che oggi vale contro la mafia e contro i reati sessuali viene esteso anche

Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, gentili colleghe senatrici, illustri colleghi senatori, intervengo per soffermarmi su un punto al quale sono molto legato, che è proprio la figura dell'agente sotto copertura che in questo dibattito è stata più volte citata, a mio modo di vedere, in maniera assolutamente inappropriata. si è descritta come fosse un marziano che atterra nel nostro ordinamento come «agente provocatore»: lo abbiano sentito dai banchi della destra, così come dai colleghi del Partito Democratico. Ebbene, penso che questa affermazione sia facilmente smentibile,

che da dodici anni ci accompagna. Quindi, la figura dell'agente sotto copertura è ben nota e sperimentata per tutti i reati per i quali oggi è operativa: stupefacenti, terrorismo, traffico d'armi, prostituzione e pedopornografia.

tanto io personalmente - lo voglio dire con orgoglio - mi sono speso insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle nel corso della scorsa legislatura, sottoscrivendo a mia prima firma il disegno di legge che cercava di promuoverla già qualche anno fa. Oggi vedo con soddisfazione che sta per diventare realtà. Perché non è un agente provocatore, egregi colleghi della destra e della cosiddetta sinistra, che ancora additate questa figura come un pericoloso sovvertimento ai principi dello Stato diritto? Innanzitutto perché vi è l'indicazione pedissequa delle norme incriminatrici dei reati contro la pubblica amministrazione. Peraltro, visto che nessuno l'ha detto, faccio notare - anche in questo caso con soddisfazione - che l'agente sotto copertura potrà essere utilizzato anche per reati di non poco conto, come l'estorsione, il sequestro di persona e l'usura; a me sembra che anche questa sia una misura da apprezzare e da favorire. Non è un agente provocatore perché, coerentemente con le statuizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché con quelle della nostra stessa Suprema corte,

promettere o dare denaro o altra utilità richiesti (richiesti) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo; o compiere attività prodromiche e strumentali. Insomma, le condotte che completano quelle già precedentemente elencate nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 non possono che riferirsi alla nuova figura dell'agente sotto copertura per i reati contro la pubblica amministrazione amministrazione e non a quelle dell'agente che cerca di corrompere il pubblico ufficiale; infatti, come è precisamente indicato, l'accordo illecito deve essere stato già concluso da altri, quindi non si provoca alcun reato. La sollecitazione da parte del pubblico ufficiale deve essere già stata formulata. Se così non fosse, in ogni caso, se questa figura di agente sotto copertura dovesse spingersi ad attività e a condotte non precisamente rientranti tra quelle indicate nella novella legislativa, evidentemente non sarebbe coperto dalla non punibilità e ne pagherebbe ogni conseguenza. Pertanto, a mio modo di vedere,

legge. Ricordo, in conclusione, che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha specificato che il compito della figura dell'agente sotto copertura è quello di disvelare un'intenzione criminosa già esistente.

si troverebbe davanti un indagato che è già pronto a commettere la violazione, anche in mancanza dello stesso intervento dell'agente di polizia giudiziaria addetto a questo tipo di attività. Pertanto, per cortesia, sgomberiamo il campo una volta per tutte dall'ipotesi che qui si stia introducendo l'agente provocatore; questo non è l'agente provocatore, che potrebbe fare ben altro e probabilmente è bene che questa figura non entri in servizio nel nostro Paese, per una serie di considerazioni delle quali condivido i timori, perché espressi con onestà intellettuale, che vengono dall'opposizione. Anch'io, signori, indosso una toga e sono sufficientemente consapevole che andiamo a toccare una materia molto delicata, che attiene all'attività della magistratura, delle forze di polizia, del diritto di difesa; tutto sacrosanto e rispettoso, ma, a mio modo di vedere, si sta incidendo sulla materia con modalità adeguate e (inutile dirlo) necessarie, dato lo stato di fatto cui il nostro Paese è ridotto a causa del fenomeno corruttivo. Vale la pena ricordare che, in aggiunta alle altre disposizioni che aumentano le pene (vedo che l'articolo 318 contemplerà una pena massima di otto anni)

Prima ancora che i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle andassero al Governo, quando eravamo opposizione e recepivamo gli *input* più ponderati e saggi sulla necessità di agire per contrastare il fenomeno corruttivo, già sapevamo in quel momento che non era solo con l'aumento delle pene che che si poteva sconfiggere e fronteggiare il fenomeno ma anche con l'utilizzo di strumenti che ne facilitassero l'emersione, perché il vero problema - come sappiamo - è quello, dato il carattere particolare del fenomeno corruttivo che vede le due parti mutualmente interessate a non far emergere l'attività l'attività criminosa. Ecco perché l'agente sotto copertura è una figura necessaria nel nostro ordinamento; ecco perché l'estensione del cosiddetto - non ho mai amato particolarmente l'espressione, però rende bene l'idea e lo sappiamo bene - Daspo per i corrotti, cioè l'estensione dei casi di interdizione in seguito a sentenza definitiva di condanna, è un altro probabilmente utile; ecco perché trovo ragionevolezza nel testo con riferimento a questa figura. Voglio spendere anche un'altra parola su un argomento che mi pare non abbia destato particolare attenzione, però l'ha

Perché è importante questa norma che estende anche ai membri delle assemblee parlamentari internazionali la punibilità per fatti di corruzione? La recente cronaca giudiziaria ha visto o vede un *ex* parlamentare coinvolto in fatti di corruzione. So che è stato assolto per il reato di riciclaggio; non so bene se è per corruzione. Il procedimento è già concluso. Parlo dell'onorevole Luca Volontè, membro del Consiglio d'Europa, e della per finanziamenti di probabile natura corruttiva provenienti da un Paese straniero interessato indirettamente alla realizzazione di quella infrastruttura che si chiama TAP. La procura di Milano si è interessata del caso e il gup ha sollevato la questione della insindacabilità e dell'immunità per la condotta di quel deputato in virtù del noto articolo 68 della Costituzione. Il pronunciamento è stato ribaltato successivamente dalla Corte di cassazione, che ha detto che, se è vero che non si può essere perseguiti per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio del proprio mandato parlamentare, questa immunità non si può estendere fino al fatto corruttivo stesso. Il voto in quel caso avveniva al Consiglio d'Europa per evitare che l'Azerbaijan ricevesse una mozione di condanna per violazione dei diritti umani e questo avrebbe comportato delle conseguenze che esulano dall'oggetto della discussione odierna, in quel caso però il consorzio promotore non avrebbe potuto attingere dai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in caso di condanna per violazione dei diritti umani.

Evidentemente quella norma comporterà che l'insindacabilità e il sacrosanto scudo della libertà di opinione e di voto dei parlamentari non si potrà estendere neanche in quella sede quando quel voto è stato frutto e oggetto di fatti di corruzione. Per questo motivo, pur essendo in discussione generale, ma non potendo intervenire domani in sede dichiarazione di voto, anticipo fin da ora il mio voto favorevole alla questione di fiducia che ha posto

turlupinare dal dito quando dietro c'è la luna. Capisco il tema, Ministro, e prendo atto del vostro punto di vista, che ovviamente non condivido. di voto del collega che mi ha preceduto mi fa capire che sto bene dall'altra parte: sono dei segnali importanti che talvolta plasticamente si manifestano anche in quest'Aula.

predicando bene, ma razzolando male. Mi viene in mente infatti che se il ministro Di Maio con la questione dei rimborsi fosse stato consigliere regionale l'avrebbero già indagato quattro volte. *(Applausi dal Gruppo quanto riguarda l'agente provocatore o sotto copertura, secondo me avete già fatto un esperimento; quando avete inviato l'avvocato Lanzalone in giro per l'Italia, prima a Livorno e poi in quel di Roma, probabilmente avete fatto una prova per vedere cosa sarebbe

perché altrimenti viene punito o cacciato; nessuno può avere un'opinione diversa. Voi vorreste che tutto il sistema nazionale, i cittadini e le imprese fossero in qualche modo bloccati

li fregate una volta e poi non più. Essi si rendono infatti conto che quando questi provvedimenti vanno avanti non portano a casa niente, nient'altro che chiacchiere e discorsi. L'unico problema è quello sulla giustizia.

prescrizione, dell'agente provocatore sotto copertura, del contratto di Governo: pian piano si dirada la nebbia ed esce il problema perché nella vostra mente - ripeto, legittimamente dal vostro punto di vista, ma noi dobbiamo opporci con tutte le nostre forze - volete tenere sotto processo chi vi infastidisce. Nel contratto di Governo avete poi scritto - e mi fa specie che gli amici della Lega, che conosco bene, lo abbiano firmato - che se per caso sei indagato o se per caso tu fossi a conoscenza che potrebbe esservi un'indagine non puoi far parte neppure del Governo.

allora staccargli la spina a questi perché, finché si parla di cosucce, va bene; quando però si parla di libertà, quando ti vengono a prendere a casa la mattina alle 6,30, poi glielo spieghi tu ai tuoi dipendenti, ai tuoi figli, a tua moglie, ai tuoi parenti, a tuo padre o a tua madre che non hai fatto nulla. Glielo spieghi tu a chi hai intorno che sei una persona onesta e perbene. Voi questa cosa non la volete:

FI-BP)*. Il signore che mi ha arrestato - e chiudo - il signor Matteo Renzi se lo è messo addirittura nel Governo a fare il Sottosegretario di Stato, perché ha fatto della carcerazione preventiva una carriera

oggi è tornato a fare il magistrato nel distretto in cui ha arrestato delle persone! Siccome poi lei è di Firenze - e ci siamo già capiti svolga il suo ruolo di controllore. Lei non è il Guardasigilli? Non guardi solo quelli; guardi cosa accade in questo Paese, guardi cosa accade nelle famiglie e nelle aziende, che sono schiacciate non da magistrati che non fanno il loro mestiere ma da una giustizia che non ha gli strumenti per andare avanti e il primo strumento glielo deve dare la politica.

signor Ministro, siamo chiamati oggi ad esprimere la fiducia su un intervento normativo, il disegno di legge anticorruzione, del quale sentiamo l'eccezionale portata, perché traduce concretamente l'impegno, innanzitutto morale, assunto nei confronti degli italiani da questo Parlamento, quello di abbattere definitivamente il tentacolare fenomeno della corruzione, mettendo in campo un'azione coordinata che si estende a raggiera, capace di colpire il fenomeno sia nel settore pubblico che in quello privato, perché la corruzione è una disonesta pratica di vita che incide, limitandola, sulla libertà e sui diritti degli italiani. I precedenti Governi ci hanno consegnato un Paese tristemente noto per l'incidenza che questo *monstrum* ha nella vita quotidiana; basti pensare che l'Italia è collocata al 54° posto nel mondo su 180 Paesi ed al 25° su 31 Paesi europei. Ma basterebbe leggere i dati dell'Autorità nazionale anticorruzione e quelli forniti dall'Osservatorio sulla corruzione nella pubblica amministrazione o semplicemente aprire un quotidiano qualsiasi, anche di cronaca locale, come ho fatto io l'altro giorno nella mia provincia, quella di Nuoro, per leggere che sono stati chiesti 15 rinvii a giudizio per sindaci e professionisti, tutti accusati di aver collaudato un sistema di malaffare che pilotava i lavori pubblici e le progettazioni, garantendo parcelle ai professionisti e voti ai politici. È partendo da questa premessa che, attraverso le modifiche del codice penale e di procedura penale, del codice civile e di alcune leggi speciali, intendiamo potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, perché sia chiaro a tutti che chi sbaglia paga e non potrà più lavorare con la pubblica amministrazione. discussione, infatti, si ampia in modo notevole l'elenco dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici "Daspo" definitivo dunque) per chi è condannato a una pena superiore ai due anni di reclusione, salvo gli effetti della riabilitazione, ma solo dopo dodici anni; non è previsto nessuno sconto, neanche per chi sceglie di patteggiare o ottiene la sospensione condizionale della pena. un inasprimento delle pene a carico del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che agisce con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, perché chi si fa corrompere deve essere punito severamente, esattamente come chi corrompe. sanzioni amministrative per una durata non inferiore a cinque anni per le società che saranno coinvolte in reati contro la pubblica amministrazione e lo *stop* anche ai faccendieri, semplici millantatori che saranno puniti per il reato di traffico di influenze illecite. La corruzione deve essere punita severamente anche nei casi meno gravi, perché comunque è un fenomeno che colpisce la parte sana della società civile, anche con effetti secondari, guastando la competizione tra le imprese, danneggiando l'economia, la meritocrazia dei cittadini. Chi sbaglia deve pagare, ma in presenza di un'autodenuncia o di una fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria viene riconosciuta, per alcuni delitti, una causa speciale di non punibilità a patto che prima delle indagini si forniscano indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili, si metta a disposizione quanto percepito, si forniscano elementi utili a individuare il beneficiario del profitto. ampliato anche l'uso delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione, riconosciute come efficace mezzo per scoprire l'attività criminosa. Anche la corruzione tra i privati è un fenomeno deplorevole. Si prevede pertanto che il delitto di corruzione tra privati e quello di istigazione alla corruzione siano siano procedibili d'ufficio. Tuttavia il problema più grande rimane quello di accertare i fatti di corruzione; per questo abbiamo individuato un valido strumento nell'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura e delle tecniche investigative speciali, già previste per i reati molto gravi dalla legge n. 146 del 2006, tutte estese alle fattispecie delittuose che configurano la corruzione. La stessa previsione di questa figura potrà essere un efficace deterrente rispetto alla commissione del reato da parte di chi non vuole correre il rischio di essere controllato e scoperto. legge prevede ancora che i detenuti per i reati di corruzione non possano accedere ai benefici premiali in sede di esecuzione della pena, a meno che non collaborino con la giustizia, così come i detenuti per i reati di mafia. Non possiamo infatti più nasconderci il fatto che i due fenomeni sono collegati: la mafia ora si occupa si occupa prevalentemente di concludere i suoi affari nell'ambito degli appalti pubblici. Concludo, signor Presidente, ricordando al PD che non è vero che in Commissione non abbiamo avuto un atteggiamento collaborativo. Mi chiedo però come si possa collaborare con una forza politica che soltanto che soltanto nel 2016 aveva firmato un emendamento secondo il quale la prescrizione cessava di operare dopo la sentenza di primo grado, emendamento che il MoVimento 5 Stelle avrebbe voluto votare,

ai miei colleghi senatori che prescrizione non significa impunità: non significa impunità per il finanziamento illecito ai partiti, per la compravendita di senatori, per il falso in bilancio all'epoca, per l'appropriazione indebita. indebita. Concludo veramente, signor Presidente, ribadendo che questo provvedimento, così come articolato, rappresenta una sfida ad ogni forma di abuso di potere rivolto contro l'interesse pubblico generale. Signor Presidente, molti colleghi sono già intervenuti su alcuni punti, ma io voglio tornare a sottolinearne alcuni, riflettendo poi sul ricorso al voto di fiducia e, quindi, anche sulla motivazione che ci porta convintamente a non votare la fiducia.

motivo di rallentamento e di confusione, perché non si capisce che ruolo abbia, si sovrappone alla magistratura ordinaria e fa grida manzoniane. Alla fine, il troppo stroppia e gli intenti, ammesso che fossero nobili, non sono stati raggiunti. a questo agente sotto copertura, a me viene anche un po' da ridere, perché quelli che ora vogliono l'agente sotto copertura sono gli stessi che hanno messo alla gogna il generale Mori perché ha cercato notizie per arrestare Totò Riina! *(Applausi dal Al telegiornale o al bar? Le cercava da quelli che gliele potevano dare e Mori ha ragione: è stato assolto tante volte e una volta condannato. Quindi, adesso, voi, che siete gli stessi, voi e i vostri giornali

a quali rischi porterà, perché un conto è combattere la corruzione e un altro è istituire figure che rischiano di istigare a dei reati. La politica, per carità, è corrosa dai fenomeni di corruzione, ma così è anche per i magistrati e le Forze di polizia: ahimè, il virus è esteso ovunque, in percentuali più o meno alte e chi lo sa se poi qualcuno non si farà tentare da un agente sotto copertura e da qualche occasione, per infangare questo o quello. Sul piano, poi, della prescrizione, vado a leggere letteralmente l'articolo 111 della Costituzione, che è stato citato anche oggi, quando abbiamo tentato di votare delle questioni pregiudiziali che avrebbero meritato il voto segreto per il rispetto della coscienza dei parlamentari, ma non è stato possibile. L'articolo 111 della Costituzione recita: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Lei ricorderà, presidente Calderoli, perché eravamo già in Parlamento, quando si è svolta questa discussione sul giusto processo e sul cambio della Costituzione. È stata una discussione importante. Oggi, come hanno detto molti colleghi, questo principio costituzionale viene calpestato, perché questo processo durerà all'infinito. Anzi, i

che lascia evaporare il 70 per cento dei processi nella fase delle indagini, perché, come ha detto oggi il presidente Bernini e come ha detto il senatore Balboni, è in quella fase investigativa che molte volte la lentezza dei magistrati fa evaporare i processi. Ebbene, allungando i termini di prescrizione all'infinito, ci sarà

gli innocenti ancor di più, perché dovranno aspettare chissà quando, ma anche i cittadini, perché la condanna immediata del colpevole è anche un ristoro della coscienza popolare. Una condanna di un colpevole che arriva dopo dieci o vent'anni non risarcisce quei cittadini che vogliono una giustizia efficace.

Penalizzate le vittime dei reati perché, quando questa sentenza mai arriverà, non avranno né la soddisfazione morale di una condanna né gli aspetti collaterali Quindi noi riteniamo assolutamente sbagliato questo provvedimento. La lotta alla corruzione va fatta invece rendendo i processi più rapidi, questo sì. Con questo provvedimento - bisogna dirlo ai cittadini - otterrete l'effetto contrario, perché credo che i processi dureranno ancora più a lungo. Nella magistratura ci sono stati grandi eroi, però c'è anche molta gente che potrebbe lavorare di più. Andate qualche pomeriggio in una procura o in un tribunale: troverete un deserto, il più delle volte. Si lavori di più in quei luoghi, per fare i processi rapidamente. Questo è ciò che serve per una giustizia esemplare e per una lotta efficace alla corruzione. Quindi, noi contestiamo dalle radici il provvedimento in esame, perché otterrà gli effetti contrari. Voi fate uso di slogan e di titoli. Non voteremo la fiducia anche per una serie di altre ragioni, cari colleghi, perché voi avete i titoli, come ha già detto qualcuno. Il decreto dignità: uno come fa a votare contro il decreto dignità? Deve essere uno indegno. Poi si è scoperto che il decreto dignità ha cancellato i posti di lavoro, 26 ogni ora. Siete degli Attila Gruppo FI-BP)*. Come ha detto qualcuno, invece che uno vale uno, unno vale unno; questo vale per voi come qualifica. Avete distrutto 26 posti di lavoro ogni ora del giorno e della notte,

L'altro decreto del ministro Bongiorno - non so come si chiamava - ha istituito un nucleo di persone che dovrebbero controllare la concretezza. Adesso 50 persone devono controllare la concretezza degli altri 50.000: un'altra pagliacciata. Chiedete la fiducia a questo Parlamento per una ragione molto chiara. Sapete perché? perché? Alla Camera il Parlamento aveva modificato il provvedimento su un punto molto delicato: il peculato. E allora, siccome ad alcuni della maggioranza non piaceva quella modifica, nata all'interno della stessa maggioranza, vi siete messi il bavaglio da soli

La fiducia è stata messa all'inizio della discussione generale; lo so che ci sono dei precedenti, ma non sono dei nobili precedenti. Chi lo ha fatto nel passato, di chiunque fosse la colpa, ha fatto male. Oggi avete soffocato il dibattito sul cambio di un principio fondamentale del diritto: la prescrizione. Vi dovete vergognare di alterare i principi fondamentali della Costituzione con il bavaglio. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non vi votiamo la fiducia anche perché state imbrogliando gli italiani. Ci accingiamo a discutere la manovra economica; ho letto poco fa che gli emendamenti arriveranno sabato. Intanto l'ecotassa c'è

Avete distrutto e smantellato le Forze armate: altro che sicurezza. Non ci sono i soldi per assunzioni adeguate nelle Forze di polizia. Le Forze armate - lo abbiamo denunciato oggi in Commissione difesa - stanno languendo e sono ridotte senza risorse in bilancio. E vedremo, dopo il ritorno di Conte dagli incontri con Juncker, quali altri tagli subirà quel settore. Avete tassato di più la casa: avete prorogato la Tasi sulla casa e non avete introdotto in modo chiaro la cedolare secca per gli affitti commerciali. Avete inventato un finto reddito di cittadinanza.

i palloncini gialli, voi dei 5 Stelle, a dire: "Onestà, onestà". Propongo un emendamento: dite a Giggino Di Maio che lo *slogan* è il seguente: "Onestà, onestà, ma non vale per papà". Urlatelo così lo *slogan*, in modo più corretto.

io non sono stupito che in quest'Aula si pronunci il nome di un condannato a dodici anni per fatti gravissimi con un'arroganza e una protervia senza limiti. limiti. Dobbiamo ricordare che il generale Mori è stato condannato da una corte d'assise di Palermo a dodici anni, per fatti gravi. È *sub iudice*, ma i fatti di cui è accusato suggerirebbero, almeno in queste Aule, di avere prudenza quando si parla di Mori, molta prudenza. L'accusa è che, mentre i servitori dello Stato, che hanno fatto la storia del nostro Paese, versavano il loro sangue, altri "si facevano sotto" - così dicevano i mafiosi - e andavano a a trattare la salvezza dei loro sodali politici, che erano nella lista di morte di Totò Riina. Questo facevano! Allora non mi stupisco, colleghi, che questo nome venga fatto adesso, in quest'Aula, da queste persone, parlando di prescrizione, perché uno di quelli che ha fondato quel partito ancora sconta una condanna a sette anni per mafia. l'altro, il signor Berlusconi...

è l'uomo più prescritto d'Italia. È vero che c'è un rapporto tra processo e prescrizione, ma è un rapporto malato che ha la radice nei vent'anni di malgoverno del nostro Paese. Paese. Dunque comprendiamo perché abbiamo assistito, in quest'Aula, all'accanimento proprio di quel partito sulla prescrizione e sulla modifica che abbiamo fatto, perché essa viene incontro alla domanda di giustizia dei cittadini di questo Paese, che non ne possono più di vedere colpevoli prescritti. *(Applausi

Dal codice penale, è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato. Sono fuori luogo tutte le parole spese per definire la prescrizione nemica di chi è innocente.

Non mi stupisce nemmeno che il PD si inalberi quando si parla di Daspo per i politici. Il Daspo va bene per i violenti dello stadio, per la povera gente, ma per i colletti bianchi non vi va bene! *(M5S)*. Dobbiamo dirle forte e chiaro che la nostra idea di giustizia non è la vostra! *(M5S)*. Quando andiamo nelle carceri e vediamo soltanto mafiosi e poveri Cristi e non i colletti bianchi che hanno devastato il nostro Paese - non li vediamo là dove dovrebbero stare - comprendiamo che dobbiamo tornare qua e fare leggi come quella che stiamo approvando oggi per mandarli in galera. Capisco, cari colleghi, che l'agente sotto copertura vi mette paura. Vi mette paura! Ma a noi e ai nostri amministratori l'agente sotto copertura non mette paura. PRESIDENTE. Senatrice Valente, vuole accompagnare fuori la senatrice Rizzotti? Anche in coppia, se volete.

un momento di maggiore genuinità per affrontare la delicatezza di questo tema, consapevole - come sono - di essere stato utente della giustizia.

Ho studiato molto e a lungo che cos'è la giustizia quando funziona, e come si presenta la giustizia quando non funziona. C'è un'immagine che ci aiuta molto di più delle urla e degli ululati che a volte si fanno per mascherare la pochezza argomentativa. Chi rappresenta la giustizia dal punto di vista immaginifico è la dea bendata. Perché la dea bendata rappresenta la giustizia, nella sua consistenza, nella sua capacità di lavoro? Deve assicurare terzietà, spersonalizzazione, genuinità, concentrazione. La prima domanda che faccio è la seguente: non siamo forse nella sessione di bilancio? Quale bisogno c'era di organizzare questa specie di spintonamento normativo in materia di giustizia penale, quivi comprendendo un ritocco impegnativo al codice di procedura e anche al codice penale? Non potevamo darci appuntamento in una seduta dedicata della Commissione per tempo e dell'Assemblea per tempo? È questo che mi fa dire, allora, che si voleva uno scalpo tematico che deve bilanciare altri scalpi che probabilmente si presume rappresentino risultati. Voglio mettere in evidenza il mio disaccordo dal punto di vista del tempo, del metodo e del merito. Parlo in nome del PD, ma parlo anche andando oltre la linea politica del PD, prendendomi qualche millimetro di autonomia espressiva. Sul piano del metodo la fiducia su questo argomento sarebbe stata bocciata dai grandi del diritto italiano. Nella mia Regione ho avuto la fortuna di studiare e di saperlo abruzzese - un personaggio, una personalità come Capograssi, il quale ci ha insegnato che anche un solo errore dal punto di vista della giustizia penale nei fatti fa passare l'ordinamento come erroneo. Dobbiamo stare attenti a queste iniziative di riforma, e mi riferisco proprio alla vicenda dell'agente provocatore. È stato detto - lo voglio precisare, avendo tanti anni di esperienza amministrativa - che è facilissimo sbagliare il superamento del confine tra lecito e illecito rispetto ad alcuni strumenti amministrativi. Ve ne cito uno: il *project financing,* nel suo essere procedura ed è legge del diritto amministrativo - è facile che assomigli all'illecito il lecito. Allora, l'agente provocatore ha un incarico, una missione destinata a fare cosa? Ad incassare quale risultato? Confacente con la funzione dello Stato o confacente con un'altra idea di efficacia dello Stato? Io ho patito - per esempio - il cattivo funzionamento di porzioni di aliquote giudiziarie che avevano l'interesse a spettacolarizzare, a organizzare l'attacco l'attacco e l'assedio. Naturalmente la giustizia mi ha dato ragione, e tante volte: 53 volte sono stato risarcito e approvato, ma non voglio personalizzare. Nella giustizia inglese i magistrati hanno le parrucche. La toga e le parrucche servono alla spersonalizzazione, al superamento dell'emotività. Per questo ho voluto chiedere la parola: noi dobbiamo evitare che una questione reale che in Italia esiste e riguarda la corruzione non determini una risposta sbagliata. C'è bisogno di rendere certe e chiare le norme. C'è bisogno di fare in modo che il personale deputato all'amministratore della giustizia sia proporzionato per i carichi di lavoro. C'è bisogno di una riforma del processo prima di fare stalattiti fare stalattiti di intervento che rischiano di rovinare l'equilibrio di cui c'è bisogno. Voglio mettere in evidenza poi un altro dato: io ho simpatia culturale per la corruzione contemplata all'interno dei rapporti tra privati, ma dobbiamo stare attenti perché, se si fa norma su un'opera pubblica che poi non nasce, non è accaduto nulla; se si fa norma che cambia il diritto penale, si fanno danni se non c'è la visione dell'insieme della conseguenza. Così come sui partiti politici c'è bisogno di fare normazione attiva prima di immaginare la patologia del suo funzionamento e finanziamento. Perché allora non darci appuntamento in un luogo che produca il meglio del discernimento, in Commissione, e poi arrivare qui senza la mannaia del voto di fiducia che uccide il confronto dialogico e dialettico. Perché? Qual è la frettolosità che determina questo livello di uccisione dell'approfondimento argomentativo e dialettico? Qual è la ragione? Non è la ragione del merito: è la ragione dello spettacolo esibire; è la ragione di incassare e intascare un argomento che poi deve essere esibito su un balcone. Ma noi abbiamo bisogno di questo, ora, in Italia? C'è bisogno di ciò? Cari colleghi senatori, io parlo da utente, consapevole però di che cosa può riservare la cattiva giustizia penale. Ho letto di recente di un sindaco di Castellaneta che ha atteso diciassette anni per vedere la fine del suo malessere personale, familiare, territoriale, di comunità politica, che ha riguardato una cattiva azione dell'iniziativa giudiziaria. C'è bisogno allora di equilibrio. C'è bisogno di fare sì che nasca il meglio di un approfondimento. Mi stava venendo in mente di dirvi: "*cum clave*" ci vorrebbe, per fare in modo che non si sbagli; per fare in modo che poi quello che insorge come risultato normativo diventi un arricchimento dell'ordinamento, e non qualcosa di strumentalizzato da una parte. C'è qualcosa della vostra visione normativa che riguarda lo Stato o è tutto di una parte sempre? Noi abbiamo l'idea della distinzione tra ordinamento, statualità, Governo, politica e maggioranza. Il diritto penale coincide con la statualità, non coincide con la parte. Non possiamo immaginare che a ogni maggioranza che interviene si dia luogo a uno strapazzamento del diritto penale, perché davvero poi, a valle, ne patiscono la collettività e l'economia. La corruzione è la rottura delle regole; è la rottura della competizione economica; è la rottura del potere per finalità particolari e questo ci accomuna nella ricerca della norma migliore. Ma non è questo il modo di procedere. Allora vi chiedo: non è possibile sospendere questo procedimento normativo e riprenderlo in un momento di tranquillità, di operosità condivisa, sapendo che poi lo lasciamo in eredità al nostro Paese, alla comunità nazionale? Non è immaginabile che su questo si faccia quello che a volte siamo riusciti a fare come - per esempio - su alcuni passaggi correttivi del Quello sforzo che stiamo sostenendo sul bilancio, per fare in modo che non tutto venga travolto dal giudizio di parte, non è possibile riservarlo a questa materia che di per sé porta delle conseguenze nella vita collettiva? Ecco, queste sono le domande con le quali voglio accompagnare la mia posizione che è emotiva, perché ho visto all'opera il diritto penale quando è spintonato. Mi sono difeso nel processo. Mi sono distanziato dalle responsabilità pubbliche. Ho atteso le sentenze. Rispetto alla prescrizione noi dobbiamo sapere che è un istituto che facilita quello che si chiama il giusto processo nella ragionevole durata del processo. Ma c'è bisogno di saperlo, però, con oggettività e laicità, capacità di ingresso nel merito. Io ho rinunciato sempre alla prescrizione, ma non avrei avuto la possibilità di attendere diciassette anni, come il sindaco di Castellaneta. Diciassette anni corrispondono alla maggiore età di un bambino che si rende poi maggiorenne. Ecco perché noi non possiamo strapazzare questi argomenti; non li possiamo rendere obolo di una collocazione politica per farsi riconoscere. Mi verrebbe da piangere su questo perché ho visto che cosa fa il Moloch, il leviatano della giustizia quando ha delle dentature sbagliate. Allora mi auguro che ci sia un soprassalto di autonomia di valutazione. Hannah Arendt diceva che c'è bisogno di autonomia del politico, ma non della figura politica, bensì della dimensione del politico quando si affrontano argomenti che durano, che perdurano, che vanno oltre la durata di una stagione.

e ha pronunciato delle parole certe, chiare. E pur essendo lontano, ho molto apprezzato, perché ho detto: «Finalmente un Ministro che forse capisce di giustizia».

non sarà mai come un suo collega di partito che ha appena parlato, il senatore Giarrusso, con il quale certamente non è possibile nemmeno scrivere una norma. norma. Quando uno non conosce il sistema di legalità, non può parlare. E non può parlare perché parla per *slogan*, per frasi da fare in una campagna elettorale, forse a Corleone dove si candidò il suo assistente, ma non certo nel nostro Parlamento. Nel nostro Parlamento si ragiona in termini di norma e se la norma ha un effetto positivo per i cittadini.

E questo oggi non è, e perché? Lei sa meglio di me, che ha un'esperienza di processi penali, come sa qualsiasi operatore di diritto che abbia esperienza nel processo penale, che più alta è la pena e il processo più lungo è, perché la pena alta porta a una prescrizione lunga e non viene mai celebrato. Non devo insegnare che tutto questo avviene dall'epoca del codice Rocco

che lei avesse già letto tutti i dati statistici del Ministero, i quali dicono che più della metà degli uffici giudiziari del nostro Paese ha una prescrizione quasi pari a zero. allora si è chiesto perché la prescrizione si concentra in alcuni uffici giudiziari, in particolare in cinque corti d'appello? E se lo ha fatto, si sarà dato una risposta e sono certo che la risposta corretta ce l'ha. La risposta è che avrebbe dovuto, prima di fare una riforma processuale di diritto sostanziale, qual è la prescrizione,

secondo i criteri della giustizia di Giarrusso, che dice che dobbiamo avere il «sospetto». Ma vi rendete conto? Dobbiamo sentire che il Daspo fa paura ai politici. A chi fa paura? A me fa paura il semplice fatto che un giurista usi la parola Daspo. A me fa paura chi non capisce di diritto e viene a parlare di cose di cui non dà nemmeno la sensazione di capire. Qualcuno ha ricordato prima Mani pulite: io c'ero a quei processi d'appello, ma da allora, signor Ministro, si è fatto quello che i magistrati dicevano? Non ad anni alterni. Qual era l'indicazione? La prevenzione. La corruzione nel nostro Paese non si scardina con pene più alte o con i processi: si scardina con la prevenzione.

per i reati contro la pubblica amministrazione significava non combattere quei reati, ma garantire maggiore impunità, e non creava deterrenza. Lei, come me, votò contro della prescrizione dopo il processo di primo grado e dopo il processo di appello, perché voleva che ci fosse un accertamento immediato della responsabilità. Solo l'accertamento nel più breve tempo possibile porta alla deterrenza.

un maggiore consenso ha portato avanti anche la prescrizione. Non credo che avrete maggiore consenso, perché i cittadini hanno difeso la Costituzione. Lei è andato in giro come me a fare comizi per difendere la Costituzione, ma non può tradirla. Non può tradirla perché, nel momento in cui introduce la pena accessoria perpetua, tradisce la Costituzione. La Costituzione vuole che ci sia la possibilità di redenzione. La funzione educativa della pena La funzione educativa della pena bisogna capirla e bisogna fare in modo che nel nostro Paese il delinquente possa redimersi e finalmente non commettere più reati. Invece no: lei vuole cristallizzare il delinquente.

Lei sa meglio di me, in quanto lo avrà studiato all'università, che già l'ergastolo è una pena grave, ma che è stata ritenuta legittima in un certo sistema.

applicare all'agente sotto copertura l'attuale legge, inserendo tutti i reati contro la pubblica amministrazione. È stato espresso un parere contrario. Perché? Devo dedurre che quella formulazione successiva, nell'attuale norma, significa che avete intenzione di rendere possibile un'interpretazione corretta o non corretta

gli amici del PD ci separano alcuni aspetti. Avete sempre detto di voler combattere la corruzione e di voler affrontare il tema, ma poi, nei fatti, non avete mai dato gli strumenti concreti affinché la corruzione fosse veramente debellata. Allo stesso modo non avete avuto il coraggio, pur dopo aver presentato un emendamento a firma Casson e Cucca nel 2016, di portare avanti le norme

che noi grillini - come ci definite - noi *parvenu* della politica siamo qui proprio per portare avanti provvedimenti come quello in Personalmente aspettavo un provvedimento serio da anni e, come me, tanti italiani; e, siccome non l'avete fatto voi, abbiamo deciso di venire noi a farlo.

tecniche investigative usate contro la criminalità organizzata come - ad esempio - l'agente sotto copertura oppure togliendo i legacci che ci sono per l'utilizzo delle intercettazioni, consentendo i cosiddetti captatori informatici e l'istituto del pentito anche in reati del genere. Insomma, si fa in modo che sia più facile far emergere la corruzione e colpirla. In secondo luogo, chi sarà condannato in primo grado non potrà farla franca contando sulla prescrizione. Infine, i partiti avranno obblighi stringenti di trasparenza e finalmente si saprà chi sono i finanziatori della politica. Questo è il nocciolo del provvedimento. Non mi bastano sei minuti per parlare di tutto ciò che contiene il provvedimento in materia di anticorruzione e per i reati contro la pubblica amministrazione. Intendiamo integrare il novero dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione oppure consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Escludiamo che la riabilitazione che - come sapete - si ottiene solo dopo tre anni dall'esecuzione della pena, possa avere effetto sulle pene accessorie perpetue. Ricordo a chi ha citato

e, quindi, è chiaro che anche in materia di prescrizione questa riforma andrà inserita in un contesto più ampio della riforma del codice del processo penale, bilanciando i diritti di rango costituzionale dell'imputato e riducendo la durata del processo. Intanto, però, di fronte a casi eclatanti di prescrizione

Concludo citando le parole pronunciate da Pertini nel 1979: «La corruzione è una nemica della Repubblica. E i corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. E dare la solidarietà, per ragioni di amicizia o di partito, significa diventare complici di questi corrotti». Bene oggi o, meglio, domani con il voto vedremo chi non avrà pietà per i corrotti e chi, invece, darà la solidarietà ai corrotti.

mi rivolgo soprattutto ai senatori del MoVimento 5 Stelle con le seguenti parole: «Se avete il coraggio, ci mettete la faccia. Venite qui in Parlamento e lo fate approvare con le regole che ha sancito la nostra Costituzione. Non venite qui e imbavagliate anche il Parlamento con l'apposizione della fiducia perché noi vogliamo semplicemente poter discutere». Sono queste le sue parole, ministro Bonafede, proponente del disegno di legge in esame, pronunciate nel giugno 2017. Ve lo ricordate, vero? MoVimento 5 Stelle, vi ricordate quando ogni fiducia gridavate e salivate sui tetti in difesa del Parlamento? Ecco che, a pochi mesi dal vostro insediamento al potere - oggi siete questo, oggi siete il potere state ripetendo gli stessi errori e le stesse forzature che per anni avete criticato quando eravate all'opposizione: totale svuotamento del senso e delle funzioni di quest'Assemblea; totale chiusura alla discussione e alle proposte delle opposizioni. Sappiamo bene perché avete chiesto la fiducia sul provvedimento: perché manca la fiducia reciproca tra gli alleati di Governo. Questo svilisce il Parlamento, ma svilisce tutti, anche voi. Ogni fiducia è un'ammissione di debolezza; il patto traballa, il contratto è carta straccia, c'è già chi chiede di cambiarlo. Allora per sopravvivere nei palazzi, per tenere il potere, per evitare una crisi che comporterebbe l'impossibilità per molti di voi di ricandidarsi - ahimè - siete disposti - e lo state dimostrando - a fare il contrario di quanto avete predicato per anni. Come si cambia per non morire. Quello che avremmo dovuto discutere oggi era un buon testo di partenza, che avremmo potuto migliorare. Ho presentato emendamenti che non saranno messi al voto con proposte che - vi assicuro - nella scorsa legislatura avreste presentato voi. Anche sulla corruzione e sul finanziamento ai partiti siete diventati più timidi e i motivi, leggendo i giornali di questi giorni, sono facili da immaginare. Per quel che mi riguarda, ho sempre considerato la lotta alla corruzione fondamentale per l'affermazione della legalità, della correttezza della pubblica amministrazione, per la prevalenza dell'interesse pubblico sugli interessi privati. È importante far emergere il fenomeno con strumenti tecnico-giuridici e mezzi investigativi più sofisticati di quelli che la legge oggi consente, in modo da colpire non soltanto le condotte di abuso di poteri pubblici, ma anche quelle ad esse strumentali o connesse. Il provvedimento in esame - gliene do atto, Ministro - introduce due importanti novità. La prima è prevedere una causa speciale di non punibilità per chi, dopo aver commesso un fatto di corruzione, prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili e restituendo le somme e le utilità date o ricevute. Un secondo rimedio è l'estensione al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, già previste dalla legge n. 146 del 2006. Bene, si sappia - ancora nessuno lo ha detto - che fino ad oggi l'Italia è stata inadempiente, sin dal 2009, rispetto all'obbligo della Convenzione di Merida di introdurre le operazioni sotto copertura in materia di corruzione. L'infiltrato - si sa - è uno che agisce sotto copertura in un'indagine giudiziaria relativa a un delitto che è già stato ideato e sta per essere commesso. L'agente infiltrato, in sostanza, si limita ad acquisire la prova di un comportamento criminale già esistente. Nel caso dei reati contro la pubblica amministrazione è stato previsto nella norma che le dazioni, le accettazioni di danaro siano in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri. Non ci possono essere dubbi, né differenti interpretazioni. È facile rendersi conto di come siano infondate - a mio avviso - le obiezioni di chi si oppone all'introduzione delle operazioni sotto copertura, facendole impropriamente coincidere con la figura dell'agente provocatore, sull'assunto che indurrebbero in tentazione persone che altrimenti non commetterebbero il reato. Nel nostro ordinamento giuridico le operazioni sotto copertura sono da tempo già previste per molti altri delitti e non solamente per i terroristi o per i mafiosi, come si è detto fino a ora. Sono previste per tanti altri reati, per reati che hanno bisogno di particolari mezzi investigativi per essere scoperti. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di rifiuti, i delitti sessuali: tutti questi reati hanno già la possibilità di essere perseguiti tramite questo strumento. Perché dunque per la corruzione non deve essere possibile? Sulla scorta di queste motivazioni, con la garanzia di specifiche modalità - non dimentichiamo che qualsiasi operazione è autorizzata e controllata dalla magistratura la raccolta di prove e non per la creazione di nuovi reati - sono favorevole all'opportunità di estendere questa tecnica investigativa ai delitti in materia di corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione. Ma se - come detto - l'elemento chiave nel combattere la corruzione consiste nella possibilità di far emergere il reato, non si deve sottovalutare l'importanza di poterlo poi perseguire efficacemente.

lo sa anche lei, Ministro - legare la discussione sulla prescrizione all'epocale, quanto non più procrastinabile, riforma del processo penale. La possibilità di mettere un punto fermo tanto atteso è un'occasione da non perdere.

e il disegno di legge in discussione prevede la definitiva sospensione e comunque la cessazione del corso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Uno dei rischi paventati è che i tempi della giustizia possano allungarsi ulteriormente, senza alcuna certezza per l'imputato di veder concluso il proprio processo in tempi la cui durata sia ragionevole, secondo l'articolo 111 della Costituzione,

il processo penale è lungo, che occorre accorciare i tempi, ma bisogna finalmente intervenire. Occorre una riforma organica del processo penale, e lei lo sa bene, signor Ministro. una procedura ipergarantista, che però si allunga a dismisura e fa allungare i tempi dei processi. Ha fatto fallire i riti alternativi, nella fondata speranza che un bravo difensore possa far ottenere

quello cioè di accorciare i tempi. Ho proposto - per esempio - l'ascolto a distanza dei testimoni, dei periti e dei consulenti; l'introduzione finalmente delle notifiche via PEC anche in sede penale (perché in sede civile sì e in sede penale no?); la lettura degli atti di polizia giudiziaria al dibattimento: tutta una serie di

la decorrenza della prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione non dalla commissione del fatto, ma dall'acquisizione della notizia del reato: sono reati che non esistono sul piano criminale perché non vengono scoperti, se non dopo anni e per caso. Non c'è nessuno che li denuncia, non c'è una vittima: l'unica vittima è la collettività. Bisogna tener conto che tali reati si scoprono dopo molto tempo e spesso si prescrivono prima ancora di arrivare al primo grado di giudizio. Sono 66.000 i reati che si prescrivono prima

non si hanno dieci anni per le indagini e, quindi, non possono prescriversi. Si prescrivono perché si scoprono e perché la data del commesso reato è il momento da cui decorre la prescrizione. Mi chiedo quindi perché non mettere tutti sullo stesso piano, in maniera tale che tutti

avremmo dovuto migliorare questo testo, signor Ministro. Da magistrato lo avrei considerato un'ottima base di partenza per un proficuo lavoro parlamentare e non cambio opinione da senatore, ancorché di opposizione. Su temi di questa rilevanza, ai quali ho legato la mia la mia intera vita processuale e professionale, non può e non deve esistere alcun calcolo politico, ma solo l'interesse generale dei cittadini. Nel mio primo giorno da senatore nella scorsa legislatura - lo sa - ho presentato un disegno di legge contro la corruzione. La logica complessiva di quel lavoro fu purtroppo recepita solo in parte, al termine di un lunghissimo *iter* parlamentare, cui ho assistito inerme da Presidente del Senato senza poter intervenire: era il mio disegno di legge. per coerenza oggi da senatore dell'opposizione avrei voluto lavorare con lei, con il suo Governo, per migliorare il testo. E lo avrei fatto con convinzione. È un'altra occasione sprecata a causa della vostra debolezza

considerando positivi alcuni aspetti del provvedimento in esame - penso all'aumento di pena e a tutta una serie di sereni intendimenti con i quali si manifesta la volontà veramente di ridurre l'impatto che ha la corruzione nel nostro Paese - tuttavia

a nostro avviso essi non rispondono a un criterio di civiltà giuridica e, quindi, di civiltà senza aggettivi. In particolare, mi dispiace che non sia presente il senatore Giarrusso, ma credo che chi parla da questi banchi - potrebbe essere chiunque del mio Gruppo - abbia pieno titolo, per la storia del nostro movimento e non solo quella personale, di dire che il tentativo di limitare la corruzione è sempre stato a destra e, insieme alla ricerca di una maggiore sicurezza per i cittadini, uno dei nostri principali obiettivi, addirittura andando oltre. Io ricordo che ci siamo persino messi un po' le mani sopra gli occhi rispetto a certi aspetti esagerati di Mani pulite, che abbiamo appoggiato forse più di quanto, con la luce che si è accesa in seguito, avrebbero meritato certe pratiche. Ma non ce ne pentiamo, perché era comunque un anelito di speranza di contrastare efficacemente la corruzione. Eppure, anche se a noi non è mai capitato di dover chiedere al nostro *leader* di fare marcia indietro per una foto con

non ci fa assolutamente specie dire che la norma sulla prescrizione è profondamente sbagliata, e ripeto profondamente sbagliata. È sbagliata, perché la *ratio* della prescrizione non sta, come un sentimento di vendetta può fare immaginare, nella volontà di colpire o non colpire il colpevole. La *ratio* della prescrizione sta nel fatto che la pena è qualcosa che lo Stato decide di comminare a un colpevole perché sia la risposta, la retribuzione, alla sua violazione della legge e anche un insegnamento alla società. Ebbene, il trascorrere del tempo in maniera eccessiva fa venir meno questa pretesa punitiva dello Stato. Ce lo hanno spiegato tutti i giuristi nella storia del diritto e lei, signor Ministro, lo sa bene. L'immaginare che, dopo il primo grado, non ci sia la prescrizione significa soprattutto incoraggiare la lentezza della definizione dei processi, perché la prima ragione la prima ragione non è quella che ci è stata detta e cioè che si scoprono tardi, la prima ragione - e non ne do colpa ai magistrati o, almeno, non solo ai magistrati - è che i processi sono lenti,

immaginare una prescrizione infinita, semmai - e abbiamo sentito anche dal presidente Grasso alcune proposte - dei rimedi per far sì che la prescrizione possa essere sospesa o che si possa consentire al processo di durare meno. La pretesa incivile, che è solo spirito di vendetta e che nulla ha a che vedere con la pretesa punitiva dello Stato,

colleghi senatori, intanto devo ringraziare il signor Ministro della sua presenza, perché lei non è un assiduo frequentatore né dell'Aula né della Commissione. Ci fa piacere vederla qui e, anzi, auspichiamo in futuro di vederla più spesso.

del Sottosegretario che ha seguito i lavori in Commissione: ho sentito la sua voce solo per l'espressione del parere conforme ai pareri sistematicamente contrari su tutti gli emendamenti.

Chi mi conosce sa che io non strumentalizzo mai nulla e che, quando parlo, ci metto sempre la faccia, in tutte le vicende che riguardano la mia attività, sia privata che pubblica. sentito strumentalizzare un emendamento che, evidentemente, non è stato approvato, facendo nome e cognome, laddove qualche altro collega, richiamando oggi l'emendamento presentato nella scorsa legislatura,

abbiamo la facoltà di pensare e tutti riusciamo anche a discernere fra quello che a noi piace e quello che a noi non piace. Al Partito Democratico quell'emendamento non piaceva e, infatti, noi, che non siamo abituati ad approvare, come fate voi, i provvedimenti solo con la forza dei numeri, voi, i provvedimenti solo con la forza dei numeri, abbiamo discusso. Sui giornali il ritiro della mia firma è stato ben riportato e, allora, conviene sempre informarsi prima di dire cose che non sono rispondenti al vero. Dico questo perché, ancora stasera, ho sentito molte parole in libertà. Abbiamo sentito che gli emendamenti non sono stati approvati perché si limitavano a chiedere la soppressione di articoli. Non è vero e qui i casi sono due: o non avete letto gli emendamenti oppure non ne avete

lo abbiate letto e abbiate compreso a cosa si riferiva e sarebbe stato bello poterne discutere in Commissione. Sarebbe stato bello sentire la vostra opinione e capire perché quegli emendamenti a voi non andavano bene. Non è sufficiente dire che volevate la corruzione con ogni mezzo: anche noi la vogliamo combattere e lo abbiamo dimostrato, con tutti i provvedimenti che sono stati approvati, spesso con l'apporto delle opposizioni. Il senatore Caliendo, che anche nella scorsa legislatura era all'opposizione, è buon testimone dei dibattiti e dei confronti che avvenivano quotidianamente in Commissione.

voi oggi state massacrando la Costituzione. L'ho già detto un'altra volta in quest'Aula: io ho giurato sulla Costituzione, ci credo, continuerò a crederci e continuerò fermamente a oppormi a questo genere di provvedimenti, che straccia i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, quella per la quale noi combattiamo qui dentro, qui dentro, mettendoci la faccia, sempre. Ma abbiamo sentito anche dell'altro. Abbiamo sentito che la prescrizione è il rifiuto della pretesa punitiva dello Stato: vedremo che risultato porterete, vedremo cosa porterete a casa introducendo questa prescrizione. Ho sentito altri stasera parlare degli avvocati. Io continuo a pensare che sia un incidente di percorso definire la classe forense come azzeccagarbugli. Debbo dire che ne ho sorriso e che non ne faccio un fatto di

nella nostra società, proprio perché ha sempre difeso quei valori di cui parlavo in precedenza, qualche volta anche a prezzo delle proprie vicende personali e qualche volta anche a prezzo della propria vita. vita. Ho sentito dire che gli avvocati spesso cercano di allungare i tempi del processo. Ma voi sapete, lo dovete sapere, che, quando un avvocato o un imputato chiedono un rinvio di qualunque genere, la prescrizione si sospende

rinviati, perché spesso e volentieri non si può procedere a effettuare le notifiche. Queste sono le cose che fanno prescrivere i processi, non l'attività degli avvocati, non quello che dite a proposito dello strumentale utilizzo del rinvio o dell'appello per cercare di allungare i processi e arrivare alla prescrizione. Vi abbiamo implorato e vi abbiamo supplicato: discutiamo di queste vicende, parliamone a viso aperto, troviamo le soluzioni. Ve l'ha detto il presidente Grasso, che, come sapete, in più di una circostanza ha manifestato posizioni che io stesso non ho condiviso, e l'ho detto in maniera aperta. Ma vi ha supplicato anche lui: proviamo a trovare le soluzioni insieme. Nulla, silenzio di tomba;

la discussione si è svolta esattamente allo stesso modo, salvo un incidente di percorso, che è stato provocato da quell'emendamento, poi fortunatamente cancellato qui al Senato, che modificava la figura del peculato per le vicende che ben conosciamo. Ora, questa è la cosa che mi preoccupa: questo atteggiamento irriguardoso delle opposizioni, irriguardoso dei principi basilari del nostro ordinamento. Lo ribadisco e ci tengo molto a dirlo: faccio l'avvocato da quasi sette lustri, quindi qualcosina nelle aule giudiziarie l'ho vista. Ma, ogni volta che faccio l'avvocato nelle aule giudiziarie, io indosso la toga e la indosso convinto, fermamente convinto, che non sia un pezzo di stoffa. L'ha detto il presidente Grasso in precedenza: non è un pezzo di stoffa. È il simbolo della difesa dei valori costituzionali, dei valori della libertà, dei valori della democrazia e della legalità

manifesto, da *spot*, per abbindolare la gente, che sarà convinta che da domani la prescrizione non opererà più. Invece continuerà ad operare più di prima, perché in questo modo, ripeto, state bloccando seriamente l'attività processuale, perché non ci sarà magistrato che penserà a quello che accade dopo il primo grado di giudizio, i processi andranno a farsi benedire e le parti civili aspetteranno una vita che vengano conclusi e definiti, se è vero, come è innegabilmente vero, che la gran gran parte dei processi si prescrive durante le indagini. E perché si prescrivono? Ancora una volta, perché non c'è personale e perché non abbiamo personale adeguato per fare le indagini in maniera corretta. Ma fortunatamente introduciamo

le pene accessorie, che restano in eterno, anche dopo la riabilitazione e, infine, introduciamo l'utilizzo sconsiderato del *trojan*. La scorsa legislatura - non si sa mai che si trovi qualche emendamento, che è stato firmato anche da me, ma che non è mai stato approvato

introduzione, perché è una cosa che interviene nella vita del privato cittadino. Non è con ogni mezzo che si combatte: si combatte sempre con la legalità e con gli strumenti democratici che il sistema Gruppo PD)*. Li abbiamo, avevate la possibilità di sfruttarli e di metterli in atto con strumenti migliori, ma avete preferito la via breve dell'imposizione di un provvedimento vergognoso, che mortifica i valori costituzionali, fondamentali nel mondo giudiziario. Ne pagherete le conseguenze, perché prima o poi i risultati verranno fuori.

profonda commozione questo pensiero, che spero unisca tutti noi in un messaggio fortemente europeista, come è sempre stato quello di Antonio.